due nuovi istituti, il pegno non possessorio e il cosiddetto patto marciano. La *ratio* di questa normativa è di semplificare e rendere più flessibile il sistema delle garanzie, facilitare l'accesso al credito delle imprese, rafforzando al contempo il sistema bancario italiano, garantendo maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore. L'impianto tradizionale delle garanzie è ormai largamente superato alla luce delle profonde trasformazioni del sistema economico. economico. L'introduzione di questi due nuovi istituti è stata segnalata da molti anni dalla dottrina più autorevole e anche da molteplici studi e rapporti internazionali. Ora, con l'introduzione del pegno non possessorio e del cosiddetto patto marciano, l'Italia è di nuovo all'avanguardia. Vorrei anticipare che nel valutare gli emendamenti nel corso delle riunioni dei lavori della Commissione finanze, i due relatori e il Governo hanno seguito la linea di preservare la semplicità del provvedimento e di evitare l'introduzione di norme che possano creare incertezza del diritto o dare luogo a contenziosi a fini meramente ostruzionistici. Arrivando all'articolo 1, che disciplina il pegno non possessorio, vorrei subito chiarire che esso consente agli imprenditori di concedere il pegno su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa senza che questi debbano subire lo spossessamento, consentendo quindi di utilizzare il bene, oggetto del pegno, per la loro attività d'impresa. Vorrei anche dire che questo sistema del pegno possessorio è molto avanzato e anche molto più moderno moderno dell'istituto della cosiddetta *sicherungsübereignung* praticato per esempio in Germania, che implica il trasferimento della proprietà del bene in capo al creditore mentre il possesso resta al debitore, perché in tal caso non vi è alcun sistema di pubblicità che garantisca anche i terzi creditori. Il nostro sistema è migliore anche di quello olandese, che prevede

Nel nostro sistema, invece, la pubblicità è assicurata con il registro dei pegni non possessori istituito presso l'Agenzia delle entrate che è già attrezzata per poter svolgere questo compito. Per questo motivo abbiamo anche respinto, in Commissione,

di specificare meglio la disciplina di valutazione degli immobili in caso di materie prime e di prodotti semilavorati poi trasformati. È il caso della concorrenza di più pegni su queste materie trasformate. Accogliendo un emendamento, abbiamo di concedere il pegno anche su crediti di terzi e precisato che il pegno può avere per oggetto beni immobili immateriali come i brevetti. Abbiamo rafforzato e semplificato l'obbligo di comunicazione in caso di escussione del pegno e disciplinato le modalità di una eventuale opposizione del debitore in caso di escussione del pegno

L'articolo 2 disciplina il patto marciano, che di per sé sarebbe già oggi lecito in base ad una ormai nota sentenza della Corte di cassazione del 2013 che ha precisato che tale patto è lecito a differenza del patto commissorio che resta vietato nell'ordinamento italiano.

Con l'introduzione dell'articolo 48-*bis* del testo unico bancario, il legislatore dà certezza giuridica a questo importante istituto e conferma l'elaborazione giurisprudenziale in materia. Vorrei precisare che tale istituito è accessibile solo a imprenditori, banche o altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti al pubblico ed è aperto, chiaramente, solo ai beni immobili. Il sistema di pubblicità è garantito con le trascrizioni nei registri immobiliari. Il vantaggio per il creditore sta nel

e chiedere il trasferimento dei beni in suo capo versando la differenza di valore stimato.

anche rispetto alle tradizionali forme di esecuzione e vendita forzata, perché non sempre, in caso di applicazione delle tradizionali modalità, il creditore riesce a realizzare un valore superiore alla stima; spesso, soprattutto nella situazione attuale di forte crisi del settore immobiliare, il ricavato di una vendita è molto minore della stima. Nel caso del patto marciano il creditore deve, invece, versare il valore stimato e non c'è alcuna possibilità di abbassamento di quel prezzo. In questo senso, il patto marciano può anche risultare vantaggioso Abbiamo tenuto conto, accogliendo una serie di emendamenti presentati da più Gruppi, delle osservazioni critiche in merito alla garanzia della *par condicio*, soprattutto rafforzando la pubblicità, con l'iscrizione nei registri immobiliari, la modifica per cui questo istituto è applicabile solo ai beni immobili e solo ai rapporti tra impresa e banche, escludendo espressamente la prima casa. Queste modalità, peraltro, erano già previste previste nel testo del decreto-legge. Abbiamo recepito le obiezioni della Commissione giustizia e di altri colleghi, che avevano ravvisato un eccessivo rigore in ordine al numero delle rate mensili e del periodo inadempimento, presupposto per il quale possa scattare la clausola del patto marciano. Abbiamo approvato una significativa modifica allungando i

prima di dover subire uno spossessamento del proprio bene immobiliare, devono passare undici mesi di inadempimento, che a noi sembra un periodo sufficientemente lungo e accettabile. Abbiamo introdotto un'altra modifica: qualora il debitore abbia già restituito l'85 per cento del capitale questi nove mesi di inadempimento devono addirittura diventare

di dover demandare alla libera contrattazione tra le parti la scelta se applicare o no il patto marciano ai finanziamenti già in essere. Siccome nessuno può essere obbligato a stipulare un contratto con una clausola di patto marciano e poiché si tratta anche di imprese e non di consumatori, pensiamo che questo possa garantire, forse, il libero gioco delle parti in campo. Abbiamo rafforzato, invece, il contraddittorio sulle stime del perito, dando facoltà al debitore di fare, entro dieci giorni, delle osservazioni, se ritiene che la stima del suo immobile fatta dal perito non sia congrua o che vi siano degli errori. In questo modo credo abbiamo rafforzato il sistema delle garanzie. Abbiamo accolto anche un emendamento che precisa che il conto dedicato sul quale debba eventualmente essere versata l'eccedenza tra il debito e il valore del bene immobile trasferito alla banca sia senza spese. Tutte le spese di questo conto devono essere accollate

al fine di facilitare la creazione di un mercato per i crediti deteriorati, si prevede l'istituzione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia, dove sono evincibili tutte le procedure fallimentari esecutive in atto ed anche tutte le situazioni di amministrazione straordinaria, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento, in modo tale che i potenziali potenziali creditori, prima di dare dei finanziamenti, possano valutare meglio la situazione economica delle imprese. Tutto questo in attuazione di un regolamento dell'Unione europea, sul modello già praticato con successo negli Stati Uniti con il cosiddetto Pacer. L'articolo 4 prevede una serie di modifiche al codice di procedura civile, per accelerare e semplificare le procedure

che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene, salvo il caso di motivi sopravvenuti o di causa non imputabile al debitore.

Abbiamo previsto, recependo un emendamento, che la riduzione del valore al 50 per cento base d'asta possa avvenire solo dopo il quarto tentativo infruttuoso di vendita e non dopo il terzo. Abbiamo precisato meglio che l'obbligo della vendita telematica di beni immobili deve avvenire dopo la messa a punto del sistema del portale delle vendite, oggi non operativo, per cui si è creata un'incertezza che abbiamo risolto con questo emendamento. Vorrei rimarcare che, anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di vendita telematica, sarà sempre possibile procedere in parallelo con il sistema tradizionale. Ritengo degna di nota anche la disciplina, che abbiamo introdotto in sede di conversione del decreto-legge, alle distribuzioni, anche parziali, del ricavato in caso di contenzioso: anche somme accantonate oggetto di controversia possono essere distribuite ai creditori, se questi creditori consegnano una fideiussione bancaria (abbiamo esteso lo stesso sistema anche al fallimento). Abbiamo precisato anche la disciplina dell'articolo 2029-*bis* per le garanzie del creditore contro cessioni del debitore di beni a titolo gratuito, per eludere il suo obbligo di adempiere. Abbiamo introdotto una

prevede l'accesso del curatore, del liquidatore e del commissario giudiziale ai dati relativi ai debitori delle procedure concorsuali, ai fini del recupero tale articolo non abbiamo apportato modifiche significative. Degno di nota è invece l'articolo 5-*bis* in cui abbiamo introdotto un nuovo elenco dei professionisti che possono provvedere

devono essere frequentati ad un decreto ministeriale. L'articolo 6 modifica alcune norme della legge fallimentare al fine di velocizzare le decisioni

sia anche significativamente importante per noi. Gli argomenti trattati all'interno di tale decreto‑legge sono cinque e vanno messi Ci sono le misure a sostegno delle imprese e per l'accelerazione del recupero dei crediti, di cui ha parlato già il senatore Zeller, e le modifiche alle procedure fallimentari, anch'esse già trattate dal mio collega.

e per coloro che hanno investito nelle obbligazioni delle banche stesse; l'ampliamento dell'operatività del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione del personale del credito e, infine, le disposizioni in materia di imposte differite attive.

aveva già svolto un'interessante indagine conoscitiva sul sistema bancario, in relazione ai meccanismi di vigilanza europei, che era arrivata a delle conclusioni nel novembre dell'anno scorso. Nel frattempo, proprio in quei giorni, si creavano situazioni di grande tensione, che vedevano l'applicazione di norme europee,

aveva fatto sì che, senza arrivare al *bail in*, che veniva recepito nel nostro ordinamento nel novembre dell'anno scorso e che sarebbe entrato in vigore dal primo gennaio del 2016, ci fosse l'applicazione della fase intermedia del *burden sharing*. di un rivolgimento totale, che rappresenta anche un momento di riflessione significativo rispetto a ciò che dovrà essere,

83 del 2015 e proprio perché c'era stata questa attenzione non si è arrivati impreparati, pur trovandosi in una situazione molto complessa che ha visto cambiare le regole del gioco mentre il gioco era in corso. Questo è

alle obbligazioni, una volta elemento di certezza e di sicurezza, e che si sono visti applicare delle norme che invece rendevano quegli investimenti molto meno sicuri, ma anche la necessità di un intervento a tutto campo che riguardasse ulteriori specificità che permettessero al sistema bancario italiano, che è un sistema bancario sano, assolutamente sano, con alcuni elementi di criticità, di poter gestire in maniera intelligente le criticità stesse.

costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. Su questo articolo 7 c'è stata da parte di diversi colleghi

di avere un'interlocuzione con il ministro Padoan, il quale già in quella sede aveva specificato che questa operazione non costituiva una vendita, ma una restituzione. L'attenzione particolare posta dai colleghi su questo tema ha fatto sì che il Governo, in sede di discussione degli emendamenti, abbia illustrato nello specifico il portato

L'articolo 8 definisce le nozioni di investitore, banca in liquidazione, nuova banca, fondo di solidarietà e fondo interbancario di tutela dei depositi. È molto importante, perché rappresenta il il perimetro alla luce del quale devono essere interpretate le norme che vengono dopo e nello specifico quelle degli articoli 9 e 10. L'articolo 9 L'articolo 9 è fondamentale, perché riguarda direttamente il tema delle procedure dei rimborsi ai clienti delle quattro banche. banche. Prima di illustrarlo penso che sia importante fare una premessa. Quello che è successo, cioè l'ipotesi di rimborso agli obbligazionisti, è una cosa *una tantum* è una cosa *una tantum* che nasce da una interlocuzione con l'Unione europea, la quale ha fissato quattro paletti che hanno rappresentato (questi invece sì) il limite dell'azione da parte della Commissione stessa. ritengo che quanto fatto dal Governo sia qualcosa di veramente significativo e comunque non più ripetibile, proprio perché rappresenta la possibilità di gestione di una fase di transizione e di tutela nei confronti di soggetti che, come dicevo prima, si sono visti cambiare le regole del gioco mentre il gioco era in corso. i paletti che sono sorti dalla interlocuzione con la dimensione europea sono: la data rispetto alla quale considerare la possibilità d'intervenire (che è quella del 12 giugno 2014), il patrimonio mobiliare di 100.000 euro, euro, il reddito lordo ai fini dell'IRPEF (che deve essere inferiore ai 35.000 euro) e l'ultimo, il termine del rimborso massimo dell'80 per cento. Come si combinano questi parametri? L'articolo 9 stabilisce che l'accesso diretto al fondo di solidarietà - e sottolineo diretto perché le fattispecie sono diverse - al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario è valido per gli investitori che siano in possesso di un patrimonio immobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro o che abbiano un reddito lordo, ai fini dell'IRPEF, nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro. è fondamentale perché è l'elemento che amplia moltissimo la possibilità di accesso diretto al fondo stesso: soggetti che abbiano acquistato strumenti finanziari di cui all'articolo 8, primo comma, lettera

e che li detenevano alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, che possono chiedere direttamente al fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e delle spese connesse alle operazioni di acquisto e della differenza positiva tra rendimento degli strumenti finanziari subordinati e rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. Viene poi specificato che la presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude la possibilità della procedura arbitrale, che nasceva dai commi da 857 a 860 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016. Parimenti, l'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esprimere le procedure dell'articolo 9, laddove questa procedura sia già stata attivata; mentre, limitatamente agli strumenti finanziari acquistati oltre il 12 giugno 2014, gli investitori possono accedere alla procedura arbitrale anche laddove abbiano fatto istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfetario e in relazione agli strumenti acquistati in data anteriore al 12 12 giugno 2014. preso atto dell'esistenza di questi paletti, abbiamo cercato di agire per rendere più facile e accessibile la procedura

ottenuto, oltretutto con la collaborazione di tutti. Preso atto che non si poteva intervenire su questi elementi, si è invece intervenuti anzitutto con una specificazione del reddito, che è passato da lordo a complessivo;

È stata eliminata la richiesta della copia di pagamento alla banca in liquidazione e del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati; è stato di fatto permesso che, per il reperimento dei documenti, le banche fossero tenute a dare copia all'investitore entro quindici giorni dalla sua richiesta. In altre parole, avevamo dei blocchi che ci impedivano di andare oltre un certo limite, ma tutto quello che era possibile fare per venire incontro al risparmiatore è stato fatto nella maniera più assoluta. Questo è stato possibile grazie al contributo di tutta la Commissione e penso anche con un po' di orgoglio da parte del Parlamento, che è riuscito a migliorare un provvedimento che apriva già prospettive assolutamente significative.

di pensare di non dovere agire per il timore che ci fosse un passo indietro e che questo venisse riconosciuto come intervento da considerarsi aiuto di Stato. Data l'eccezionalità dell'intervento, che nasceva dalla necessità di gestire una fase di transizione che ha visto delle persone essere soccombenti e danneggiate dall'introduzione delle nuove norme, la possibilità di individuare dei parametri che venissero loro incontro ha visto la necessità di incontrarsi in modo significativo con il livello europeo. Il limite di 100 milioni, introdotto nella legge di stabilità, è stato invece abolito ed ha portato al 30 giugno il termine per l'emanazione dei decreti del Ministro dell'economia. Questo è un tema importante e delicato perché,

dall'altra, invece, c'è la possibilità del ricorso arbitrale. È però giusto che il cittadino sia posto nella condizione di poter scegliere se utilizzare uno strumento o l'altro, e senza l'emanazione di tali decreti ci si trova in una situazione monca, perché da una parte si sa esattamente qual è la procedura, ma dall'altra non si ha la possibilità di scegliere, perché non si sa quali siano i criteri che verranno adottati per la procedura arbitrale. È pertanto importante procedere in questo senso in tempi strettissimi da parte del Ministero.

di far sì che il versamento avvenga non solo da parte della consolidante, ma anche in qualità di consolidati; è stato inoltre presentato un emendamento sostitutivo dei relatori, che ha reso più facilmente interpretabile ed applicabile la norma stessa anche per un problema di sovrapposizione di tempi. L'articolo 12 invece introduce una deroga, per gli anni 2016-2017 con riferimento al personale del credito, della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterale. Il tema dell'articolo 12 è delicato, perché avremmo voluto fare di più. Innanzitutto, avremmo voluto poter intervenire anche nei confronti delle banche di credito cooperativo e avremmo voluto ampliare le possibilità con una serie di emendamenti che erano stati presentati, ma purtroppo vi è stato un vincolo molto forte nei rilievi operati dalla Ragioneria generale dello Stato. Abbiamo pertanto deciso, come Commissione, che si interverrà con l'approvazione di un ordine del giorno unitario per cercare di sviluppare e approfondire nuovamente questi temi in modo da dare una risposta a una questione piuttosto delicata. L'articolo 13 invece agisce in materia di copertura finanziaria. Questo è il veloce prospetto del decreto Ribadisco concludendo che tale provvedimento non va considerato in quanto tale, ma come un'ulteriore perla di una collana che sta affrontando la questione del sistema bancario italiano - ribadisco, un sistema bancario sano sano - che non ha mai ricevuto aiuti di Stato, a differenza di quello che è successo in altre realtà. La Germania, che adesso è così rigida - permettetemi questa considerazione - ha dato alle proprie banche 237 miliardi. Noi, in un interessante prospetto, abbiamo visto che i soldi erogati, sono stati poi restituiti, permettendo peraltro un piccolo guadagno per lo Stato di 100 milioni. troppe volte vediamo emergere nei *mass media* solo una serie di elementi negativi. È giusto dire che noi ci stiamo occupando con attenzione di questo tema, ma, poiché il substrato su cui stiamo operando è fertile, ci auguriamo possa rimettere in moto quel meccanismo di ripresa di cui il nostro Paese ha sicuramente bisogno. Questo decreto-legge, anche con gli apporti dati dal Parlamento, credo possa rappresentare

Fino ad oggi, viste le proposte di riforma in ballo, la funzione legislativa spetta collettivamente alle Camere e questo dovrebbe essere un principio.

per alcuni provvedimenti, quando anche le opposizioni sono coinvolte nella giusta misura, la trattazione di un argomento non è eccessivamente dilatata e può avvenire con tempi che permettono un vero esame e approfondimento della materia.

Non si può continuare ad attaccare norme e modificare articolati senza tenere conto dell'apparato organico e sistematico delle norme.

Le leggi sono quelle che inquadrano l'insieme di un processo. Intorno a quel processo, non ruotano solo il magistrato e l'avvocato, ma anche i cittadini.

vogliamo parlare di questo provvedimento, in particolare per chi sta fuori da quest'Aula, perché si renda conto di cosa stiamo votando. Voglio parlare a quei cittadini radunati qui fuori e che stanno manifestando. Siamo davanti all'ennesimo decreto salva banche: sì, salva banche. Il relatore lo ha definito una perla. E non poteva proprio dare una definizione migliore. È l'ennesima perla in questa collana di perle che sono i vari decreti salva banche approvati in questi mesi. In realtà questo è un cavallo di Troia, perché, dietro all'accattivante titolo che reca «Norme a favore degli investitori in banche in liquidazione», esso nasconde trappole. Una vera e propria truffa semantica, al pari della truffa perpetrata alle spalle dei risparmiatori. Con questo decreto-legge il Governo, di fatto, si preoccupa di favorire la riscossione dei crediti da parte delle banche, introducendo procedure sempre più veloci, che si rivelano potenzialmente letali per le imprese. E solo marginalmente, come vero e proprio fumo negli occhi, introduce anche delle norme per il risarcimento dei risparmiatori truffati. Infatti, prima di tutela dei risparmiatori ha aspettato per poter trovare il modo migliore per salvare anche le banche. Risparmiatori truffati - ripeto: truffati - e non investitori audaci e spregiudicati come qualcuno ha avuto il coraggio di definirli. Vogliamo ricordare da chi sono stati truffati? Sono 130.000 risparmiatori che hanno perso i propri risparmi custoditi in azioni, obbligazioni subordinate di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara, Cassa di risparmio di Chieti. E sono solo le ultime quattro in ordine temporale rispetto alle precedenti; il primo nome, Banca Etruria, ormai tristemente famoso, in quanto legato al padre del Ministro per i rapporti con il parlamento, Maria Elena Boschi. Sono risparmiatori che hanno visto andare in fumo i loro risparmi, ingannati una volta e oggi ancora una volta ingannati da questo Governo che aveva promesso di tutelarli: il Governo Renzi-Boschi, il governo di Banca Etruria. Etruria. Siamo di fronte al solito decreto-cavallo di Troia: dietro all'apparente intento di provvedere alla salvaguardia dei risparmiatori truffati dalle banche, già salvati *in extremis* sempre da questo Governo, prima le banche e poi i risparmiatori, il decreto-legge che, anziché tutelare i risparmiatori, tendono a tutelare le banche e a permettere un più agevole recupero dei crediti sempre da parte delle stesse; ma poche sono le norme volte a consentire un agevole recupero dei crediti da parte dei risparmiatori e a incentivare la disponibilità del credito da parte degli istituti bancari. Signori, questo Paese soffre. Soffre quando soffrono le piccole e medie imprese che ne sono l'anima, soffre quando le piccole e medie imprese chiudono per una scarsa disponibilità economica. Soffre quando un'impresa chiude perché non è riuscita a investire per diventare più competitiva nel mercato. Diventare più competitiva a volte significa investire denaro nuovo, significa potersi permettere macchinari nuovi e nuovi beni strumentali, e per farlo, purtroppo, oggi serve il finanziamento delle banche. Banche che quel finanziamento non lo danno. Per renderlo più facile, per riportare le banche a fare il loro dovere, la loro *mission*, la loro funzione principale, non si interviene sulle banche, non si impongono criteri tali da rendere il credito da parte delle banche obbligatorio, da spingerle a farlo, disincentivando le banche che non svolgono questa funzione in modo adeguato. No, assolutamente. Lo si fa, al contrario, incentivandole. Alle banche va sempre riconosciuto un incentivo, vanno premiate se fanno quello che in teoria dovrebbe essere il loro dovere. E come vengono incentivate? Introducendo una serie di norme e codicilli che permettono di

Si potrebbe far funzionare meglio la giustizia, renderla più celere, permettere ai giudici di avere le risorse necessarie per rispondere alle numerose richieste in tempi ragionevoli e con la certezza della verità. E invece no; anche in questo caso si tenta la via stragiudiziale, si cerca di far sì che le banche diventino giudici di se stesse e dei propri debitori, innescando meccanismi perversi di ricatto e soggezione. È così che entrano in gioco le norme del pegno non possessorio che permette alle imprese di mettere a garanzia del debito bancario un bene mobiliare riguardante l'attività produttiva. Attenzione: «permette alle imprese», perché questa la modalità con cui voi presentate queste norme. È una possibilità in linea teorica, ma di fatto aumenta a dismisura il potere contrattuale delle banche, essendo le imprese spesso a corto di liquidità e finanziamenti a causa della situazione di crisi e quindi costrette a inserire nel contratto con la banca la nuova disciplina, La cosa comica è il modo in cui viene presentato, come un'opportunità, una possibilità, la solita truffa semantica, per dire che da domani tu, impresa, avrai uno strumento in più, ma in realtà quello strumento in più è che potrai impegnarti i beni di famiglia, quelli dell'azienda, come una volta si faceva al banco dei pegni. Bello strumento! La banca non rischia mai niente, la banca presta soldi come se non facesse parte di questo sistema Paese, come se non risentisse direttamente della crisi. Man mano che le aziende chiudono, chiudono i conti correnti, chiudono le linee di credito e chiudono le banche. È una conseguenza naturale. Voglio ricordare le parole di Nick Hanauer, uomo di affari americano: «Mentre persone come voi e me prosperano oltre i sogni di ogni plutocrate nella storia, il resto del Paese - il 99,9 per cento - resta molto indietro e arretra. Il divario fra quelli che hanno e quelli che non hanno peggiora sempre di più. Io guadagno all'anno 1.000 volte l'americano medio, ma non compro mille volte più roba. La mia famiglia negli ultimi anni ha comprato tre automobili, non 3.000. Ho acquistato qualche paio di pantaloni e qualche camicia all'anno, come molti altri americani. Ho comprato due paia dei migliori pantaloni di lana, ma non avrei potuto acquistarne 1.000. invece messo via il mio denaro *extra*, là dove non fa molto bene al mio Paese. Se i 9.000.000 di dollari di Hanauer in più dei 10.000.000 di guadagni annuali fossero andati a 9.000 famiglie invece che a lui, sarebbero stati pompati di nuovo nell'economia attraverso il consumo e avrebbero creato più occupazione. Questi soldi stanno invece nei conti bancari di Hanauer o investiti in società che non hanno abbastanza clienti potenziali a cui vendere. C'è poi il famoso passaggio automatico della proprietà dei beni immobiliari delle imprese alla banca, esclusione del bene adibito ad abitazione principale. Attenzione, so già che il Governo farà apparire ciò come una grande vittoria, dicendo che ha impedito che le banche possano appropriarsi dell'abitazione principale, nascondendo però che, dietro questo, possono appropriarsi di tutto il resto in caso di ritardi nel pagamento. Viene saltata la procedura giudiziaria davanti al tribunale, al tribunale, che ha così il solo compito di nominare un perito per stimare il valore dell'immobile. Chi tutela il debitore da un'eventuale truffa della banca? Chi lo tutela da un calcolo errato di interessi o rate laddove decide di non pagare perché, appunto, ritiene che ci sia un errore o una truffa? Anche in questo caso si tratta, in linea puramente teorica, di una scelta facoltativa dell'impresa, ma come possiamo immaginare che si tratti di una scelta libera quando chi ha il coltello dalla parte del manico è sempre la banca? Chi ricorre al credito di una banca è perché ne ha bisogno e sappiamo bene che le banche non danno soldi a chi non mette davanti un valore corrispondente e nessuna banca eroga un prestito o apre una linea di fido se non dietro la garanzia di un bene che possa essere prontamente acquisito. Magari sarà una forma di differente agevolazione negli interessi e avremo i crediti agevolati (cioè uguali a quelli di adesso) e i crediti ordinari (cioè più cari di quelli di adesso) nell'uno o nell'altro caso. Si prevede anche che il credito delle banche disciplinato nell'articolo in esame prevalga giuridicamente su tutti gli altri crediti, compresi quelli dei fornitori dell'impresa e dello Stato, ad esempio le imposte. ha la precedenza su tutti gli altri creditori. Ma quale banca non si getterà a pesce su questa nuova forma di strozzinaggio? Diamole infatti il nome che si merita: strozzinaggio. Dicono che la norma non sia retroattiva, ma il dare la possibilità di inserire questo patto nei contratti di credito già in essere la rende di fatto retroattiva.

questa riforma, che non so come definire se non come un ennesimo regalo alle banche. Siamo dinanzi all'ennesimo decreto-legge, all'ennesima fiducia, all'ennesimo svilimento del Parlamento, all'annullamento del dibattito e della discussione, alla volontà di rendere la Costituzione carta straccia.

Voi ve ne fregate di noi e dei cittadini che rappresentiamo e proseguite sempre con la stessa arroganza e sbruffoneria che il vostro capo vi ha insegnato.

non formale. Quello in esame è un provvedimento estremamente complesso su cui - voi colleghi lo potete testimoniare - abbiamo cercato, per quanto possibile, di dare il nostro contributo.

È un provvedimento molto opaco, che si basa su degli errori compiuti nel passato, ancora inemendati. È un provvedimento che presenta elementi di criticità sotto il profilo formale, procedurale e sostanziale. Non voglio essere troppo burocratica. Noi abbiamo presentato una questione con un contenuto molto espanso. Abbiamo voluto entrare anche nel merito perché, mai come in questo provvedimento, la forma è sostanza e la sostanza è forma. è forma. Avendo i canonici dieci minuti per illustrare tutte le perplessità costituzionali che abbiamo nei confronti di questo decreto-legge,

l'altro ad ogni controllo di questo Parlamento perché purtroppo la maggioranza vince e noi dell'opposizione possiamo denunciare le patologie, ma non possiamo fermare la corsa del treno anticostituzionale, rappresentato da questo provvedimento sulla base di criteri di disomogeneità che sono denunciati dallo stesso titolo. È infatti il titolo che ci racconta che all'interno di questi provvedimenti c'è la violazione costituzionale. È lo stesso titolo che ci racconta che non esistono quella necessità e quella urgenza previste previste dall'articolo 77 che, evidentemente, il presidente Renzi ritiene di poter modificare per via consuetudinaria. A forza di fare decreti-legge totalmente sprovvisti dei presupposti di necessità ed urgenza, pensa che prima o poi l'articolo 77 si considererà cambiato dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Sta facendo giurisprudenza. In realtà, noi non lo abbiamo capito, ma il suo obiettivo è quello di fare giurisprudenza. Sta, però, a noi denunciare la patologia insita in tutto questo. Credetemi, è un'ironia molto amara quella che stiamo facendo. stiamo facendo. Si tratta di un provvedimento particolarmente infelice sotto questo profilo, perché noi abbiamo un ulteriore elemento di grande criticità che si innesta sull'incostituzionalità, dato dalla modalità brutale, e sottolineo di predisposizione delle leggi. Modalità brutale, sciatta e inefficace. Anche questa volta facciamo norme strappate strappate da una finta emergenza e innestate su un corpo di norme che deve essere stabile, chiaro, assolutamente trasparente ed inequivoco, per dare ai suoi utenti, tutti i cittadini, e ai suoi interpreti, la certezza del diritto. Noi, con un decreto-legge disomogeneo, cambiamo insieme, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, il codice civile, il codice di procedura civile e la legge fallimentare. Ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo? In ogni provvedimento, peraltro d'urgenza, in ogni decreto-legge totalmente sprovvisto dei requisiti di necessità e urgenza, sta un pezzettino di cambiamento dei testi fondamentali per la vita democratica e per la certezza del diritto di questa Repubblica. Colleghi, è alquanto inquietante, anche perché queste modifiche, su cui ora entrerò nel merito, oltre ad essere assolutamente inopportune, incostituzionali e creare e creare un ulteriore elemento di confusione nel corpo normale e naturale di queste discipline sono anche profondamente inique.

nella parte più delicata di questo provvedimento che il presidente Marino ha cercato di giustificare attraverso i quattro paletti dell'Europa. Collega Marino, lei ed io insieme abbiamo avuto a che fare con l'Europa nella scorsa legislatura, e sappiamo che l'Europa rappresenta certe volte un velo di Maya che, le assicuro, i risparmiatori traditi dalle quattro banche decotte non vedono l'ora di squarciare. Non credo che i risparmiatori traditi - poi passerò alle modalità di risarcimento parziali, insufficienti e assolutamente discriminatorie che prevede questo decreto - saranno contenti di sapere che l'Europa ha previsto un criterio temporale per il loro soddisfacimento o dei parametri di reddito e di rendita che - per carità, riconosco alla Commissione di aver cercato di dilatare quanto possibile - ma che rimangono assolutamente insoddisfacenti. Colleghi, Presidente, presidente Marino, perché il rimborso forfetario? Avete questo riflesso vagale, lo avete fatto anche con le pensioni, per la mancata indicizzazione delle pensioni per due anni. Voi decidete e addirittura lo chiamate *bonus*, come se faceste pure una cortesia ai risparmiatori, risarciti

Grazie, patologia che si innesta su un'altra patologia. Noi vi abbiamo detto e ve lo ripetiamo a proposito di questo provvedimento: non facciamo leggi *spot*, non facciamo leggi di apparente soddisfacimento di alcune istanze, che ritenete non rinviabili e che poi ci rimbalzano in faccia con una una violenza straordinaria. È successo per gli 80 euro, e sarà un dramma perché gli 80 euro dovranno essere restituiti da persone che li hanno già spesi e che hanno un reddito addirittura inferiore ad 8.000 euro. E lo stesso accadrà a questi risparmiatori perché, colleghi, non facciamo finta di non sapere che tutte queste belle intenzioni non hanno ancora un canale di attuazione. Il presidente Marino lo diceva prima, con molta delicatezza, ma questo famoso Fondo di solidarietà cui si dovrà attingere per risarcire, in maniera - ripeto - assolutamente parziale, iniqua e discriminatoria, solo una porzione minimale dei risparmiatori delle quattro banche - lasciando fuori peraltro gli altri risparmiatori di tutte le banche popolari e di credito cooperativo di cui si stanno rivelando adesso le truffe che non sono ricomprese in questo provvedimento - è un canale ancora ancora chiuso perché ci vogliono i decreti attuativi. Ancora una volta abbiamo davanti un provvedimento ad efficacia differita, totalmente in controtendenza rispetto allo spirito del decreto-legge, anche se ormai abbiamo capito che per Renzi il decreto-legge è una categoria dello spirito non un modo di legiferare dotato, purtroppo, di caratteristiche di normazione primaria. Però, ripeto, non esistono ancora i modi per questo risarcimento. Concludo, Presidente, perché

arbitrale per la regolamentazione della quale ci si riferisce alla legge di stabilità, è ancora totalmente priva di contenuti, come privo di contenuti e di fondi è il Fondo di solidarietà attraverso cui dovranno essere risarciti questi risparmiatori. Parliamo, ancora una volta, del nulla, di modalità che avrebbero potuto essere attuate, poste in essere mesi fa, quando il Governo avrebbe dovuto farlo non con uno strumento come il decreto-legge ma con un atto di normazione secondaria, con un decreto ministeriale. Se si fosse voluto, si sarebbe potuto farlo potuto farlo in maniera corretta, in tempi congrui e per un equo ed efficace soddisfacimento dei risparmiatori. Ancora una volta, colleghi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che racconta tante cose, promette tante cose ma minaccia di mantenerne molto ma molto poche. Per tutti questi motivi e per tanti altri ancora che abbiamo indicato in maniera molto più analitica nella nostra pregiudiziale, chiediamo che il percorso di questo provvedimento si fermi qui.

Signora Presidente, questo provvedimento è l'ennesimo intervento normativo di riforma del settore bancario con lo strumento del decreto-legge. Secondo il disegno costituzionale - ogni volta insistiamo su questo elemento - i decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati a operare immediatamente allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare sopravvenute e urgenti necessità, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Da ciò, quindi, discende immediatamente l'inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare riforme di sistema, quale quella contemplata in questo provvedimento e anche in altri che abbiamo esaminato recentemente. Non è, quindi, lo strumento del decreto-legge che può intervenire su materie come queste, che incidono direttamente sul diritto sostanziale e processuale, anche con rilevanti ricadute sul sistema socioeconomico. Le modifiche al codice bancario e al codice di procedura civile, Grazie,

Alcune disposizioni, infatti, sono destinate ad entrare in vigore solo dopo l'adozione di regolamenti di attuazione ed altre non introducono alcunché di innovativo ma solo adempimenti stringenti in capo ai soggetti che operano in ambito esecutivo, individuale e concorsuale. Tra l'altro - se entro più specificamente nel merito di alcune disposizioni,

le misure contenute negli articoli relativi al sistema delle garanzie, all'accelerazione del recupero crediti e alla riduzione dei tempi delle procedure esecutive, non sono finalizzate a sostenere le imprese o i cittadini, bensì, introducendo istituti e strumenti nuovi, ad avvantaggiare e rafforzare unicamente le banche, che avranno, tra l'altro, ancora maggiore facilità per conciliare i loro unici interessi. i requisiti restrittivi per l'accesso al Fondo di solidarietà previsti dall'articolo 9, ovvero le scelte del Governo di circoscrivere il beneficio solo a coloro in possesso di un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro

presso altri istituti bancari di beneficiare del rimborso forfettario, introducendo una distinzione giuridica tra clienti privati delle quattro banche che hanno acquistato sul mercato secondario e privati investitori che hanno acquistato presso altri istituti ed includere nel conteggio del patrimonio mobiliare dell'investitore gli strumenti finanziari subordinati azzerati per evitare gravi distorsioni a danno di chi detiene quote importanti di tali strumenti finanziari per cento) sono solo alcune delle numerose norme discriminatorie presenti nel provvedimento che escludono dal rimborso automatico intere categorie di risparmiatori ledendo in maniera rilevante il principio parimenti le disposizioni in materia di espropriazione forzata, in particolare la liberazione dell'immobile pignorato senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario il trasferimento dell'immobile tramite l'attivazione del patto marciano svolgendosi unicamente su impulso del creditore, senza la presenza del giudice non offrono sufficienti garanzie al debitore e in mancanza di contrappesi vi è il reale rischio che le banche possano imporre la nuova forma di garanzia per concedere il finanziamento all'imprenditore, con la possibilità, in caso di inadempienza del debitore, di diventare proprietari del bene violano il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione; l'articolo 4 incidendo in modo rilevante sulle procedure delle aste giudiziarie impone una vera e propria svendita del patrimonio privato violando l'articolo 42, comma 2, a tutela della proprietà privata. Nello specifico viene previsto che il tribunale può disporre massimo tre esperimenti di vendita, ognuno con un ribasso di un quarto rispetto al precedente prezzo. Qualora tutti dovessero andare deserti, il magistrato potrà disporre una quarta asta, facoltativa, riducendo addirittura il prezzo dell'immobile fino al cinquanta per cento. Ad aggravare l'impatto negativo contribuisce l'efficacia retroattiva della norma che si applica anche a tutti i pignoramenti immobiliari anteriore alla riforma ed ancora in corso, e per quelli in cui sono svolti tre esperimenti d'asta, che quindi possono essere chiusi anticipatamente al ribasso dal giudice; dal giudice; la norma relativa alla procedura arbitrale, alternativa alla richiesta di rimborso forfettario, non chiarendo le modalità in cui si svolgerà l'arbitrato, non consente ai risparmiatori di decidere quale procedura intraprendere e non consente al risparmiatore di accedere alla procedura di arbitrato qualora la procedura per ottenere l'indennizzo forfettario non si concluda per mancanza dei requisiti o per l'impossibilità di reperire la documentazione richiesta e soprattutto non prevede esplicitamente che l'accesso alle due procedure, di rimborso forfettario e arbitrato, non precluda l'avvio o la prosecuzione di azioni risarcitorie, civili o penali, nei confronti delle «Nuove banche» o di altri soggetti attentando a

Signora Presidente, nonostante la buona stampa che accompagna ancora il Governo Renzi, a differenza di qualche tempo fa...

il testo che stiamo esaminando può essere annoverato nell'elenco delle interpretazioni fornite dal Governo sulle sue azioni, che ricevono regolari smentite, più o meno diplomatiche, anche nei più importanti consessi istituzionali. L'ultima in ordine di tempo arriva dalla Banca d'Italia, che riduce le stime di crescita e raffredda le aspettative per un aumento dell'inflazione; lo stesso ha fatto l'OCSE, che ha aggiunto anche la previsione di un rallentamento del *trend* occupazionale,

ci siamo trovati di fronte a provvedimenti generici - e questo decreto-legge è uno di quelli - dalla prosa il più delle volte involuta, pieni di errori e a volte di orrori di varia natura, dal banale refuso al reiterato rinvio a norme non più vigenti, non più vigenti, provvedimenti che un'istituzione degna di questo nome non dovrebbe nemmeno accettare di discutere. Questo Parlamento si è ridotto a fare l'ufficio legislativo del Governo,

la forma diventa drammaticamente sostanza, come ha detto la collega senatrice Bernini, e il provvedimento che esaminiamo sta proprio dentro questo *vulnus*, per cui si interviene con un decreto-legge in un ambito in tra diritti compressi e innovazioni, stiamo cambiando la faccia dell'economia del Paese. Nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri che approvò il decreto-legge in esame, il presidente Renzi lo ha salutato come il provvedimento che avrebbe risolto in maniera definitiva i problemi del sistema bancario nazionale: un sistema sano, a detta di tutti, ma che evidentemente proprio tanto sano non doveva essere, se quattro banche, come quelle che sono state ampiamente citate, tutte nel Centro Italia, hanno posto all'attenzione di tutti noi il fatto che, probabilmente, nella regolarità delle loro attività,

Perché in realtà il decreto-legge, articolato nelle tre parti che sono già state ampiamente citate soprattutto dai relatori che mi hanno preceduto, è tutt'altro che sistematico. che sistematico. Nelle prime due parti, quelle più direttamente rivolte alla soluzione dei problemi degli istituti di credito, il testo governativo si caratterizza per la frammentarietà e lo scarso approfondimento delle dinamiche e delle conseguenze immediate e future delle disposizioni che contiene. A cosa mi riferisco, signora Presidente?

un sostegno all'annoso problema del sistema bancario, delle sofferenze, dei crediti incagliati e di quelle situazioni che, all'indomani della sventurata e irresponsabile approvazione del *bail in* da parte del Parlamento, compresa quest'Assemblea, è è emersa all'attenzione di tutti. È esploso il bubbone di quelle sofferenze che dentro i bilanci delle banche costituivano un drammatico appesantimento che impediva poi, nell'ambito della vigilanza europea, alle nostre banche di poter continuare a svolgere

altro che un intervento marginale e secondo noi ancora farraginoso e pletorico sulla ridefinizione dei due istituti già utilizzati nella pratica e nelle attuali procedure espropriative. Essa determina un intervento squilibrato, apparentemente in favore delle banche, ma solo apparentemente, perché in realtà nemmeno alle banche servirà questo provvedimento, che di sicuro non servirà a contemperare le legittime ragioni di tutte le parti è già stato detto, chi si occuperà dell'equilibrio corretto tra creditore, debitore e altri creditori a vario titolo? Perché ci preoccupiamo solo di di risolvere una parte del problema, quando questa era l'occasione per intervenire, soprattutto in testi così complessi e delicati come quelli della procedura civile, a favore di tutte

una visione meramente finanziaria dei cosiddetti *non performing loan*, che sono certamente un tema finanziario, ma se inseriti in una visione veicolata da chi opera sui mercati internazionali (quelli che frequentano i salotti delle banche, dove le azioni si pesano e non si contano) attraverso questa visione macro dei problemi è abituato a standardizzare. Questo lo fa anche la BCE e anche quel sistema di vigilanza che ha inteso assumere uno *standard* che non contempla minimamente realtà economiche e finanziarie

non pensare unicamente allo *spread* o a margini operativi per risolvere questo problema, ma avere una visione più di dettaglio, perché a questo serve l'analisi che è stata fatta dal lavoro della Commissione, peraltro pregevole. il senso delle proposte che abbiamo presentato si muoveva nella consapevolezza che banche e imprenditori, banche e imprese, sono parte di un unico sistema, vitale per l'economia nel suo insieme, che non può rinascere privilegiando privilegiando una parte a scapito dell'altra; è solo responsabilizzando tutte le parti in gioco che possiamo davvero cambiare il verso, in modo che non sia solo un *hashtag* o un tormentone, ma sia una realtà seria seria e concreta a favore delle nostre aziende. Vorrei concludere questo mio intervento in discussione generale ricordando che nel buon lavoro della Commissione molta attenzione è stata posta a migliorare il testo, ma non ne è stata posta

che questo provvedimento ci auguriamo possa risolvere, ma che invece temiamo non risolverà.

un pericolo gravissimo che sta per essere introdotto nel nostro ordinamento a danno delle imprese e a preciso e sfacciato vantaggio delle banche e degli istituti finanziari. Vediamo di spiegare in poche parole in cosa consiste questo patto, la cui ammissibilità è certamente stata già dichiarata dagli organismi giurisprudenziali italiani e anche dalla dogmatica, ma che, per le condizioni in cui sta per essere introdotto, ci porta assolutamente nel campo del killeraggio delle imprese. Si tratta di poter trasferire la proprietà o il diritto reale di un bene immobile direttamente in favore del creditore senza passare attraverso le procedure esecutive note, quelle che vedono il normale *iter* dell'atto di precetto, del pignoramento, della vendita e della possibilità del debitore esecutato di potersi difendere tutte le volte in cui il credito azionato sia contestabile. Nel caso di specie, per quanto riguarda le banche, chi ha conoscenza dei tribunali sa benissimo che il contenzioso giudiziario relativo alla quantificazione dei crediti delle banche banche è molto frequente. Mi riferisco alle note questioni relative all'anatocismo bancario, alle clausole illegittime contenute nei contratti di mutuo, agli interessi anche di tipo usurario che sono conteggiati, con procedimenti anche penali che spesso nascono in danno delle banche e dei loro rappresentanti legali. Qui il punto, cari colleghi, è che, introducendo nel testo unico bancario il nuovo articolo 48-*bis*, stiamo facendo entrare - come ha detto il collega Crimi - un cavallo di Troia, ed è bene che gli imprenditori italiani sappiano sin d'ora a quale rischio vanno incontro nel momento in cui chiederanno un finanziamento, un mutuo alle banche. Ma soprattutto - ahinoi - anche coloro che hanno già in corso un finanziamento e un mutuo potranno cadere in questa che può essere una trappola mortale per le imprese. Diciamolo chiaramente: l'avverarsi della condizione che permetterà alle banche di apprendere direttamente il bene immobile messo a garanzia si verifica con il solo mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive. in Commissione finanze, aderendo in minima parte alle sollecitazioni del Movimento 5 Stelle e anche di altre opposizioni, è stata parzialmente modificata la norma, prevedendo che il ritardo nel pagamento di ogni singola rata non sia più di sei mesi (come oggi stabilito nel testo unico bancario) ma di nove mesi. mesi. Questo evidentemente è un pannicello caldo che non metterà le imprese al riparo dal rischio di perdere la disponibilità dei beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione del debitore, del coniuge e dei più stretti congiunti. Per fortuna, almeno ancora c'è questo limite, ma certamente non servirà a liberare

La giustificazione del relatore Zeller, secondo la quale comunque occorre una sottoscrizione volontaria per far operare questo patto, in realtà è una giustificazione vuota, nulla, perché sappiamo benissimo, e sfidiamo chiunque a dimostrare il contrario, che oggi un istituto bancario che ha in corso un

oltre al volere introdurre questo patto marciano, è renderlo applicabile ai finanziamenti in corso: questo porterà migliaia di imprenditori italiani a mettersi un cappio intorno al collo perché, nel caso

che le banche adesso, allontanandosi da quella che dovrebbe essere la loro funzione storica, istituzionale ed economica, stiano creando società immobiliari

creditizio funzionale è una risorsa ed è una necessità per fare andare avanti l'economia del Paese e le imprese. Ma le condizioni in cui il sistema bancario opera in Italia credo siano note a tutti e quindi, richiamando quanto il relatore ha esposto nella sua relazione con riferimento al patto marciano, che già esiste in altri Paesi europei come la Germania e l'Olanda per cui non c'è rischio a introdurlo anche in Italia, sfido il relatore o chiunque altro a dimostrare che la situazione normativa e la tutela dei correntisti, dei risparmiatori e degli imprenditori che accedono al finanziamento bancario nel nostro Paese sia uguale a quella dei Paesi citati. Così non è, e la cronaca quotidiana ci dà notizia di quanto il quadro normativo a a tutela del risparmiatori e dei correntisti lasci molto a desiderare. Per di più è previsto che questo Per di più è previsto che questo patto valga anche per le procedure esecutive pendenti, quindi siamo veramente alla follia. Nelle procedure esecutive in corso, la banca che si sarà fatta firmare questo patto creditorio abbandonerà la procedura esecutiva per la prensione diretta del bene. Tutto questo a discapito delle ragioni del debitore, delle imprese in questo caso, tutte le volte in cui ha motivo di contestare il credito. Non a caso oggi, nelle procedure esecutive immobiliari, nelle cancellerie delle sezioni commerciali dei tribunali, ai delegati alla vendita, cioè a coloro che quantificano il credito delle banche, sono inviate circolari per specificare i criteri, per evitare che le banche, come fanno e cercano di fare molto spesso, carichino il loro credito di interessi o di altre voci non dovute. Tutto questo sparirà. il dover ricorrere ancora una volta al decreto-legge, l'avere infilato questa normativa nell'ambito di un farlocco sistema di risarcimento per i risparmiatori truffati dalle quattro banche è l'ennesimo sfregio che questa maggioranza e questo Governo vogliono imporre,

con il taglio dei nostri stipendi, e vederle con il cappio al collo per questa normativa vergognosa è qualcosa contro la quale ci opporremo in ogni maniera. Presidente, colleghi, penso che questo sia l'ennesimo provvedimento che interviene in materia di credito in questa legislatura,

finanziario e alla tutela di percorsi di arricchimento sul possesso del capitale, piuttosto che

dello sviluppo del nostro Paese in Europa e per affrontare i gravi problemi di natura sociale che subisce

che la struttura del provvedimento tende a salvaguardare gli istituti di credito e le banche, che non possono essere e non sono il fine del sistema economico, bensì uno degli strumenti per sorreggere il nostro sistema economico. Io che vengo da sinistra, non sono un grande appassionato dell'economia di mercato, che affida alle regole della della relazione economica tra soggetti il destino di un'economia; sono più perché si ritorni a fare una programmazione economica e perché sia sia rilanciato l'intervento dello Stato e della comunità, perché una comunità esiste e sta in condizioni di benessere se pensa a se stessa e l'esclusione progressiva

sviluppano percorsi di accumulazione parassitaria che rendono molto più complicato lo lo sviluppo dell'economia e il mantenimento di livelli di benessere sociale nel nostro Paese, in Europa e in Occidente. Suggerisco a tutti la lettura dell'ultimo libretto che scrisse Galbraith prima di morire: «L'economia della truffa». Ci siamo affidati ai maghi della cosiddetta finanza, che divorano anche loro gran parte delle risorse che si producono e sono superpagati per mantenere alti i livelli di redditività del capitale, cancellando possibilmente e devastando il sistema produttivo.

una garanzia sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, per continuare a esercitare l'attività d'impresa e avvalersi del credito per poter sviluppare la propria azienda. La realtà è che, in un sistema che è soffocante per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, questo diventa uno strumento attraverso il quale si rende ostaggio l'impresa. Il sistema finanziario, il sistema del credito e le banche così come le stiamo producendo hanno hanno poco interesse a svolgere una delle principali funzioni per le quali sono nati, cioè raccogliere il risparmio e destinarlo ad investimenti, certo garantiti, ma funzionali allo sviluppo economico. La banca oggi ha una preoccupazione, quella di mantenere il più possibile nelle proprie casse la propria liquidità per farne oggetto di speculazione finanziaria, perseguendo l'arricchimento

capacità manageriali nel settore produttivo nel quale si decide di investire ed è sottoposta a difficoltà che derivano spesso da andamenti, anche di mercato, che si decidono in altre parti del mondo, molto difficilmente controllabili e in mano a soggetti che sfuggono totalmente anche alle regole dei singoli Paesi. Ebbene, siccome questa è la dinamica, il risultato è che anche ciò che apparirebbe utile, ai fini dell'accesso al credito, diventa uno strumento di consegna come come ostaggio al sistema del credito e della finanza, perché insieme alla costituzione del pegno non possessorio c'è un sistema degli interventi di recupero dei crediti che assume una caratteristica veramente rischiosa. Le dinamiche con le quali si concludono le aste giudiziarie e le procedure connesse a quelle aste giudiziarie hanno la logica di chi vuole approfittare del fallimento, mettendo lo stesso istituto di credito

nella condizione di approfittare e di speculare sul fallimento. E lo fa attraverso la partecipazione all'asta giudiziaria per conto terzi,

preferito - e non rinunciamo a pensare che si possa fare - adottare finalmente una normativa quadro sul credito, che consenta a tutti, alle imprese, ai cittadini, oltre che agli operatori di quel settore, di capire dove stiamo andando e quali sono i rischi di questo sistema per poter funzionare a beneficio della comunità. *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che giunge oggi in Assemblea si colloca all'interno di un complesso percorso di riforma del settore creditizio italiano, che si inserisce nel più ampio processo in atto a livello europeo. Permettetemi di farvi dono di un episodio presentatosi alla mia persona pochi giorni fa e, per essere più chiari, vi voglio parlare di una frase che da alcuni giorni è oggetto dei miei pensieri: «È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli» XVII)*. È una parola essenziale per comprendere il rapporto di Gesù con la ricchezza. L'immagine è forte, paradossale, com'è nello stile semitico. Tra la ricchezza e il Regno di Dio c'è incompatibilità ed è inutile voler annacquare un insegnamento che più volte ritroviamo nella predicazione di Gesù, quando dirà, ad esempio, che non si può servire Dio e Mammona (cioè la ricchezza). O quando sembra chiedere al giovane ricco rinunce impossibili all'uomo, ma non a Dio.

Mi dispiace contraddirla, Presidente, ma è argomento proprio della discussione. Che cosa condanna allora Gesù? Non certamente i beni di questa terra in sé, ma chi è attaccato ad essi. E perché? È chiaro: perché tutto appartiene a Dio e il ricco invece si comporta come se le ricchezze fossero sue. Il fatto è che le ricchezze prendono facilmente nel cuore umano il posto di Dio e accecano e facilitano ogni vizio. Paolo, l'apostolo, scriveva: «Coloro che vogliono arricchire, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al denaro, infatti, è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori». Quale allora l'atteggiamento di chi possiede? Occorre che egli abbia il cuore libero, totalmente aperto a Dio, che si senta amministratore dei suoi beni e sappia, come ha detto Giovanni Paolo II, che sopra di essi grava un'ipoteca sociale. I beni di questa terra, non essendo un male per se stessi, non è il caso di disprezzarli, ma bisogna usarli bene. Non la mano, ma il cuore deve stare lontano da essi. Si tratta di saperli utilizzare per il bene degli altri. Chi è ricco lo è per gli altri. «Io ho scelto Dio solo, nessunissima altra cosa» e sono certo che quando apparirò davanti al Dio dei nostri padri, il suo figlio e nostro fratello Gesù non mi dirà: «È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel Regno dei Cieli». E per voi, miei amati fratelli, banchieri, bancari, parlamentari, religiosi, economisti, imprenditori e commercianti, spero che le vostre sorde orecchie non sentano l'assordante grido nel deserto del coerede di Dio e nostro signore Gesù Cristo dirvi: «È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel Regno dei Cieli»! Ma adesso ritorniamo al disegno di legge, oggetto del mio intervento. Vi stavo parlando del provvedimento recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione». Il testo si prefigge l'obiettivo di accelerare il recupero del credito a tutela di chi concede finanziamenti. Come sapete, ho già affrontato il problema più e più volte in passato, schierandomi dalla parte di tutti quei cittadini e consumatori vessati da tassi di interesse fuori controllo e da indebiti bancari di varia natura. A maggior ragione oggi, mi sento di fare una riflessione profonda perché pare che la situazione non sia destinata a migliorare. Nella Bibbia si legge: «Il ricco domina sul povero e chi riceve prestiti è schiavo del suo creditore». una realtà che è rimasta tristemente immutata nei secoli anzi, che forse è stata ulteriormente aggravata da una bramosia di ricchezza che ha portato a creare delle vere e proprie mostruosità in tema di economia mondiale. Sto parlando di signoraggio, ossia il reddito derivante dall'emissione di moneta, quel flusso di moneta derivante dalla differenza tra il valore reale e quello commerciale delle banconote stampate. plusvalenza viene sottratta al popolo italiano in virtù della perdita della sovranità monetaria, attuata da una *lobby* di affaristi

promuovendo la riscossione dei crediti tramite procedure più veloci, ma potenzialmente letali per le imprese, prevedendo anche un parziale pasticcio, perché non è equo il risarcimento per i risparmiatori truffati. Con il pegno non possessorio di cui all'articolo 1 del decreto-legge, che mette a garanzia il bene mobiliare dell'impresa (attività, mezzi, strumenti, attrezzature e adesso mi dicono anche crediti), si aumenta di fatto in modo spropositato il potere contrattuale del soggetto già più forte, ossia l'istituto creditizio, costringendo di fatto le imprese ad accettare l'inserimento nel contratto della nuova disciplina,

non ricevere l'erogazione del credito. passeranno direttamente nella proprietà della banche in caso di inadempienza nel pagamento dopo un certo numero di rate non pagate in un determinato lasso di tempo. Un lasso di tempo che in Commissione è stato anche allungato, ma le rate restano tre, anche non consecutive, e quindi ben lontane dalle sette rate che erano considerate necessarie per vantare il credito previsto dalla il credito della banca magicamente prevale giuridicamente su tutti gli altri creditori in caso di fallimento, sia i fornitori che i lavoratori e anche lo Stato con le imposte. Agli articoli dall'8 al 10 si disciplina il risarcimento per i risparmiatori truffati nel salvataggio delle quattro banche popolari tramite il tristemente famoso decreto salva banche: grande ammissione di colpa del Governo. Questo risarcimento sarà però solo per l'80 per cento e solo per risparmiatori con reddito complessivo

requisiti rigidi, inconcepibili e limitati tra l'altro solo a chi ha acquisito obbligazioni subordinate prima del 12 giugno 2014, ossia prima della pubblicazione del *bail in,* che poi con questo provvedimento non ha alcun rapporto, anche il *bail in* è diventato esecutivo nel dicembre. Non si capiscono quindi i motivi di questa data. Tutti gli altri si dovranno avvalere dell'arbitrato. si verranno a creare inevitabilmente paradossi di rimborsi milionari e di mancati rimborsi per redditi di poche migliaia di euro di differenza e non si eviteranno ricorsi, con danni generali per tutti, per gli imprenditori e per le banche. In conclusione, ripetendo cose già dette più volte e ribadite anche in Commissione da auditi di un certo rilievo, ma che noi riteniamo sempre importante ribadire, le banche hanno abdicato da lungo tempo alla loro funzione originaria di sostegno all'economia reale, atta a fornire il diritto al credito, che è costituzionalmente sancito, agli individui, alle famiglie e alle aziende, e al dovere di accompagnare e sostenere nel percorso imprese, piccole e grandi, iniziative, progetti e *start-up*. Le banche, come noto, concentrano come noto, concentrano ormai quasi tutte le loro attività in funzioni esclusivamente speculative in ambito finanziario, perseguite troppo spesso con del rischio dei risparmiatori e con conseguenti danni enormi sull'economia del Paese. Questa situazione ha avuto negli anni riflessi fortemente negativi sull'economia reale e questo non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma lo dicono gli analisti del settore della grande crisi economica che ci attanaglia ormai da decenni. Come se non bastasse, le banche troppo spesso si dedicano a funzioni concorrenziali. Concorrenza certamente sleale proprio nel mondo imprenditoriale che dovrebbero sostenere, occupandosi di funzioni direttamente commerciali, quali vendite di di beni ed erogazione di servizi (adesso si stanno organizzando al meglio per il grande patrimonio immobiliare che gli pioverà addosso). La banca deve tornare al suo ruolo sociale, deve rinsaldare la sua attività attività con il tessuto produttivo concreto. È necessario che le banche siano spinte a rischiare a fianco degli imprenditori e tornare così a produrre ricchezza reale per tutti, creando imprese concrete e tangibili che producano beni, servizi e lavoro. la Lega Nord non condivide né il metodo con cui si sta portando avanti questo provvedimento, né il merito e i contenuti di questo testo, che introduce dei cambiamenti secondo noi molto rilevanti nel rapporto tra banche e debitori, imprese e famiglie. Ci sembra che i temi e l'importanza di questo provvedimento siano trattati con molta leggerezza, trascuratezza, e poca attenzione persino dagli organi di informazione. Passano spesso da quest'Aula provvedimenti di rilevanza molto relativa

uno per uno, votandoli. Ogniqualvolta viene portato avanti, invece, un provvedimento rilevante che ha incidenza sulla vita reale dei cittadini in difficoltà, quasi sempre la procedura adottata da questo Governo e da questa maggioranza è la stessa, decreto-legge è inaccettabile. Si cerca ogni volta di eliminare il disturbo provocato dall'attività parlamentare per espressa volontà del Presidente del Consiglio. È una procedura assolutamente antidemocratica autoritaria che precede quanto avverrà se passerà la riforma costituzionale promossa da Renzi. Bisogna eliminare il disturbo provocato dal voto degli elettori e dall'attività parlamentare in Assemblea: questi sono i due capisaldi dell'attività legislativa così come la intende il Presidente del Consiglio; un esercizio del potere senza che la rappresentanza dei cittadini possa incidere. È vero, in Commissione è avvenuta una discussione approfondita, però dobbiamo notare due cose. In primo luogo, l'accoglimento degli emendamenti è, a nostro avviso, superficiale. Sono stati accolti emendamenti che correggono errori evidenti del decreto-legge, e su quelli evidentemente anche la maggioranza ha dovuto chinare il capo e fare ammenda; c'erano poi emendamenti che avrebbero modificato in modo sostanziale il provvedimento su cui invece la maggioranza si è limitata ad approvare alcuni emendamenti di facciata che danno una risposta assolutamente parziale e insufficiente ad aspetti di grande rilevanza.

Siamo disposti, purché non si arrivi alla fiducia, a ritirare gran parte degli emendamenti che abbiamo ripresentato in Assemblea e a mantenerne solo 30 relativi ai temi che avevamo sottolineato anche in Commissione

Sappiamo che per quanto riguarda il patto marciano la norma prevede che dopo tre rate non pagate e un tempo che è stato alzato da sei a nove mesi si mette in moto un procedimento assolutamente rapido di fronte al quale il cittadino non ha possibilità di difendersi, finalizzato a fargli perdere le sue proprietà

un debitore andrà in banca e chiederà di rivedere le proprie istanze e le proprie situazioni debitorie, o chiederà nuovi prestiti. Ogniqualvolta che lo farà, è evidente che la banca avrà una posizione di forza per chiedere, a fronte di tale ridiscussione, l'introduzione del patto marciano.

È evidente che vengono tolte tutte le garanzie che avevano i cittadini per difendersi dall'aggressività di questi meccanismi che possono metterli sul lastrico. Cambiano sostanzialmente i rapporti di forza tra le banche e i cittadini e tra le banche e le imprese a favore delle banche. Abbiamo poi presentato una serie di emendamenti all'articolo 9, perché i requisiti che avete adottato per accedere al risarcimento sono molto stretti.

tutelate i risparmiatori truffati, quando nella realtà volete togliere dal tavolo un problema politico con una risposta assolutamente inadeguata e parziale.

può riconoscere l'indennizzo (obbligazioni sottoscritte prima del 12 giugno 2014); tutta la documentazione che deve produrre il cittadino truffato; le procedure complesse attraverso le quali ottenere questi indennizzi. Sono risposte assolutamente inadeguate, che dimostrano una sola volontà del Governo, quella che ha portato avanti anche con il decreto salva banche: tutelare gli interessi dei forti e di abbandonare a se stessi diritti dei cittadini truffati. Questo è il vostro indirizzo e questo è l'indirizzo del provvedimento, che noi contestiamo e di fronte al quale manifestiamo tutta la nostra contrarietà. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi in discussione, come questo Governo ci ha abituato, è totalmente discrezionale, è un palliativo. Il Governo toglie il veleno da una ferita, tutela solo una parte senza guardare al quadro d'insieme. Non è stata, infatti, studiata una soluzione valida per tutti, che offra un'effettiva tutela, anche nel lungo periodo. Da un testo che entra nei tema delle esecuzioni ci si aspetterebbe un intervento normativo che, ferma la tutela dei creditori, finalmente impedisca la svendita dei beni degli

Si parla di un abbattimento dei prezzi che possa superare anche il 70 per cento del valore di mercato. Nemmeno i creditori sono soddisfatti di tali svendite restando quasi sempre a bocca asciutta. Nel migliore dei casi solo le banche ottengono qualcosa dalle aste. Questo sarebbe stato l'unico intervento davvero urgente in materia esecutiva, eppure il Governo riesce nell'impresa di peggiorare una normativa già catastrofica, vessando ancora di più i debitori e lasciando i creditori, ad eccezione delle banche, largamente insoddisfatti. Per quanto riguarda, poi, le disposizioni relative agli investitori delle banche in liquidazione, quello che mi preme maggiormente sottolineare è la situazione in cui sono incappati gli investitori della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Dalla lettura degli articoli 8 e successivi del provvedimento in discussione, infatti, è possibile comprendere come le misure urgenti da adottare a favore degli investitori da applicare in presenza di determinati presupposti risultino esperibili solo nei confronti degli investitori delle seguenti banche: Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti. Ebbene gli azionisti della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca resteranno fuori e non potranno conseguire alcun indennizzo. Si tratta di un folto numero di azionisti, che forse sarebbe meglio definire vittime. Infatti anche Veneto Banca, come Banca popolare di Vicenza, è costretta ad azzerare il valore delle azioni, per quanto entrambe si dicano disponibili ad andare in conciliazione con tutti i loro clienti possessori di azioni (visto che ormai tali azioni sono così svalutate ed invendibili, tutto ciò non sembra altro che un tentativo per chiudere la vicenda a poco prezzo, senza garantire un giusto e adeguato risarcimento ai risparmiatori coinvolti). Si tratta poi di conciliazioni che, nella maggior parte dei casi, partono con una lettera di richiesta di risarcimento e si concludono in un nulla di fatto. *e-mail* è piena di richieste di aiuto da parte di risparmiatori, che sottolineano il fatto che Veneto Banca ha venduto queste azioni senza informare i consumatori dei possibili rischi, abbassandone poi il valore dell'80-90 per cento rispetto a pochi mesi prima e rendendo di fatto nulla la possibilità di rivenderle. Si tratta di famiglie, lavoratori, piccole aziende e associazioni che si sono fidate di banche in cui si investiva da generazioni; persone che hanno risparmiato una vita adesso si ritrovano con niente mano. Ma questo Stato non dovrebbe difendere il risparmio, così come sancito dall'articolo 47 della Costituzione? Nel dicembre 2015, ad esempio, Veneto Banca aveva fissato il prezzo di recesso delle azioni a 7,30 euro, obbligando di fatto gli azionisti che avessero voluto liberarsi delle azioni a perdere l'81 per cento del valore di ogni azione e generando una violazione dei diritti e degli interessi dei consumatori, stabiliti dal codice del consumo e dalla normativa dei settori bancario e finanziario. Gli azionisti di queste banche sono posti in una tale situazione di inferiorità da sembrare surreale. Infatti le due banche non solo hanno tagliato il prezzo, ma impediscono ufficialmente agli azionisti di avvalersi del diritto di recesso. Le perdite scaturite sono superiori ai 7 miliardi di euro: una cifra maggiore, quindi, a quella delle altre quattro banche messe assieme citate nel presente disegno di legge. È inaccettabile che debbano essere i risparmiatori a dover pagare le difficoltà degli istituti bancari. Per salvare le banche, infatti, potrebbe scattare il meccanismo del *bail in*, per cui proprio i possessori di azioni e obbligazioni sarebbero obbligati a mettere i soldi di tasca propria per tenere a galla l'istituto di credito. I piccoli risparmiatori che fanno la fila davanti agli sportelli delle associazioni di tutela dei consumatori sono tantissimi e la speranza che possa esserci per loro un risarcimento delle perdite subite è sempre più remota. Non si tiene conto di tutti quei risparmiatori che erano convinti di investire i risparmi di una vita, con l'assicurazione che il rischio sarebbe stato bassissimo, più che altro a causa delle comunicazioni false e fuorvianti dei consigli di amministrazione attualmente oggetto di indagini, che, a ben vedere, non sono mai stati oggetto di controlli incisivi da parte degli organi di controllo del sistema bancario. Come spesso accade, a rimetterci sono i lavoratori, le famiglie e quei piccoli imprenditori che già coraggiosamente tentavano di farsi strada in un periodo di profonda recessione. Concludo augurandomi che si vorrà tener conto di una soluzione a più ampio raggio, che miri effettivamente a far sì che non ci sia un crollo totale della fiducia dei risparmiatori nell'intero sistema bancario, coinvolgendo, in casi del genere, gli azionisti e gli obbligazionisti per tentare una soluzione condivisa, affinché non vengano più estromessi dalla BCE. Soprattutto, mi auguro che si voglia estendere le procedure di rimborso anche agli azionisti delle banche popolari venete, onde evitare una crisi economica che peserà che peserà per decenni sull'economia e sulla società veneta e non solo.

il tema del risarcimento ai risparmiatori truffati e il tema dell'offerta che viene fatta alle imprese. Riguardo al discorso dei risparmiatori, abbiamo un risarcimento dovuto,

si vedono risarciti come per una specie di grazia, che viene loro da un Governo che però non li ha saputi tutelare precedentemente.

è che non si è voluto tener conto di un ordine del giorno che chiedeva quantomeno di considerare tale situazione. Il risarcimento a questi risparmiatori va posto in essere al cento

alle imprese si concede la possibilità di prendere prestiti per comprare attrezzature e poi si requisiscono gli immobili. Gli immobili non fanno credito e nessuno ha voluto considerare che tale situazione di acquisizione di immobili diventa un ulteriore vantaggio per le banche in fallimento. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il provvedimento in esame viene emanato con modalità di urgenza e ancora una volta assistiamo al ricorso alla questione

I provvedimenti del Governo che abbiamo visto finora (e non sono stati pochi) non hanno portato alcuna soluzione alla crisi del sistema bancario. È vero, al contrario, che le regole europee sulla vigilanza e il sistema di vigilanza stesso hanno ricreato, anche se con ritardo, un nuovo quadro di certezze. Va detto che la Banca d'Italia è stata intempestiva su molti dei provvedimenti adottati e questa intempestività la spinge ora a considerare favorevolmente alcuni provvedimenti adottati dal Governo. In realtà, se si fosse intervenuti prima nei casi delle quattro piccole banche in amministrazione straordinaria, si sarebbe evitato anche il decreto-legge odierno per indennizzare gli investitori truffati; tuttavia, quello che secondo me è più importante e che più ci sta a cuore è che probabilmente avremmo evitato queste truffe. Vorrei preliminarmente preliminarmente sottolineare, ricordandolo a me e a tutti i colleghi, che gli indennizzi dovuti agli inconsapevoli investitori delle quattro piccole banche andranno sicuramente a pesare sulla fiscalità generale.

il recupero dei crediti. In realtà si aiutano le banche a cedere sul mercato i propri crediti deteriorati e si agevolano altresì gli istituti che, dopo averli acquistati, li andranno a recuperare, forzatamente e con procedure più facili, anche mediante procedure stragiudiziali. Sarà infatti possibile agire sia sui beni immobili che su quelli mobili, attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento, come tanti hanno ricordato questa mattina, dell'istituto del pegno non possessorio. Sono questi i beni che quasi sempre costituiscono gli strumenti principali per l'attività di una impresa o di un professionista. Si crea in questo modo una nuova gerarchia dei creditori: i primi creditori non saranno i soggetti più deboli (dipendenti e fornitori), ma diventeranno gli istituti di credito. In realtà, in Italia le banche non sono arrivate allo stato di amministrazione straordinaria a causa dei crediti deteriorati, ma, nella maggior parte dei casi, per operazioni finanziarie fraudolente. Il deterioramento dei crediti è stata solo una conseguenza della pessima gestione, riconducibile a gruppi manageriali di scarsa qualità professionale, etica e morale. È il caso del Monte dei Paschi di Siena, della Carige, della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, quattro banche che erano grandi e in alcuni casi prestigiose. Nel loro piccolo anche la Banca Popolare dell'Etruria, Carife, Cassa di risparmio di Chieti e Banca delle Marche hanno dimostrato, nel migliore dei casi, di possedere un *management* inadeguato che le ha malgestite. La cosa più angosciante è il fatto che mentre la vigilanza faceva anche piccoli passi per controllarle, le banche malgestite erano legate tra loro da una sorta di *fil rouge*, tanto che per assurdo quando la Banca Etruria aveva già dimostrato evidenti segni di difficoltà, l'unica offerta di integrazione arrivata era stata, ironia della sorte, della Banca popolare di Vicenza, che pure di problemi ne aveva e assai ben più gravi. In realtà è il mercato che alla fine regola ogni cosa e al momento stiamo assistendo a un livello di speculazione altissimo sui nostri istituti di credito quotati, che li sta costringendo a continui aumenti di capitale, anche laddove questi siano dotati di patrimoni importanti. Vi sono al momento banche che posseggono un patrimonio netto pari a cinque volte la propria capitalizzazione di borsa: questo significa che i corsi azionari sono con tutta evidenza soggetti a speculazioni di breve periodo. Dall'altro lato va rilevato che entrano nel capitale delle banche italiane anche fondi di investimento di lungo periodo. Questo è certamente un segnale importante del riconoscimento del valore intrinseco degli istituti di credito italiani. di credito italiani. Da una parte, quindi, l'azione della BCE, dall'altra quella dei nuovi criteri per la vigilanza bancaria hanno creato le condizioni per un sistema bancario più forte - si può dire - nonostante gli interventi poco risolutivi in questo campo del Governo. In realtà quello che manca ed è sinora mancato (posto che in natura nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma) è un provvedimento che vada a recuperare le risorse sottratte fraudolentemente alle banche da chi le gestiva; ma soprattutto manca ancora un quadro di fiducia, di maggiori certezze normative, regolamentari e di controllo che faccia crescere il volume di risorse che le banche destinano all'economia reale. È questo il grave problema di cui dovremmo occuparci, e questa dovrebbe essere la nostra prima attenzione perché senza questa attenzione e senza questa volontà di occuparci del problema, rischiamo di non agganciare questa fase ciclica di crescita economica. Signora Presidente, il mio intervento si concentrerà sostanzialmente sugli articoli 8 e 9, ovvero quelli riguardanti misure in favore degli investitori delle banche in liquidazione. Il lavoro parlamentare di questi giorni ha ulteriormente migliorato il testo del decreto-legge, che - lo dico con nettezza - ha rappresentato già un rilevante, significativo passo in avanti rispetto alla misura legge di stabilità, ottenendo un risultato capace di risarcire al cento per cento tutti coloro che sono stati truffati. Ciò attraverso il superamento del tetto dei 100 milioni per il fondo attivato con la legge di stabilità, perché tutti coloro che sono stati truffati devono essere risarciti, e lo saranno attraverso le due modalità previste: l'indennizzo automatico e l'arbitrato. Sottolineo che con la previsione dell'automatismo, e dei requisiti requisiti per accedere ad esso, si è fatta una scelta che ha guardato con grande attenzione alle fasce più deboli. Nel passaggio parlamentare, che ha costituito davvero un lavoro significativo e proficuo, anche il riferimento al reddito di 35.000 euro, uno dei due requisiti per accedere all'automatismo, è stato migliorato stabilendo che il reddito cui si fa riferimento non è quello lordo ma quello complessivo, così come definito dall'articolo 3 del TUIR, con la conseguenza importante di allargare la platea di coloro che possono accedere all'automatismo. Si tratta davvero di un elemento fondamentale che, insieme alle tante altre modifiche che sono state apportate, migliora il provvedimento, grazie anche ad un lavoro importante

correttezza e trasparenza, potrà ricorrere all'arbitrato ottenendo il 100 per cento. A tal proposito tengo a precisare quanto sia importante il contenuto dell'articolo 10, che prevede che entro il 30 giugno sia adottato dal Governo il decreto attuativo riguardante le procedure dell'arbitrato. Ciò

all'azione continua, pressante, propositiva e tenace del Governo, a partire dal Presidente del Consiglio Renzi al ministro Padoan, che abbiamo convinto l'Europa. Ricordate, colleghi, la cautela con cui, in punta di piedi, il ministro Padoan ha dovuto cercare a dicembre

tutti i cittadini, della cui truffa non è responsabile il Governo o questo Parlamento. Voglio ribadire quali sono stati i risultati importanti di questo percorso parlamentare. Dentro i quattro paletti categorici dell'Europa (i 35.000 euro, i 100.000 euro, la data del 12

Un altro elemento di novità è l'allungamento dei tempi per la presentazione delle istanze al fondo: si passa infatti dai quattro mesi ai sei mesi. Ed ancora di grande rilevanza è la facilitazione per la documentazione che l'investitore dovrà allegare all'istanza; tale documentazione dovrà essere fornita dalla banca entro quindici giorni dalla richiesta. Tengo anche a sottolineare che è stata chiarita dagli uffici la questione della cointestazione, che era un elemento di grande preoccupazione.

l'obbligo di vigilanza ai fini del contenimento del rischio, della stabilità patrimoniale e della sana e prudente gestione da parte degli intermediari, la Consob ha invece, anche sulla base della legge

Mi domando allora perché la Consob, anche dopo l'agosto 2013 quando è entrato in vigore il *burden sharing* (ma anche dopo) ha continuato a permettere che fossero emesse obbligazioni subordinate da collocare al dettaglio, la cui rischiosità era dissimulata ed il cui rendimento, che andava tra il 4 e il 5 per cento, era di poco superiore agli altri titoli pubblici. Mi chiedo inoltre: perché la Consob ha tolto dai prospetti di vendita gli scenari probabilistici? Vegas ha detto più volte che questo era vietato dall'Europa, ma non è così: l'Europa invita invece ad inserire nei prospetti di vendita gli scenari probabilistici.

di queste indagini. Ciò che ha portato la Banca Etruria ad essere liquidata è stata proprio la *mala gestio*, la scelleratezza con cui sono stati fatti prestiti e investimenti totalmente slegati dal territorio, frutto di gestioni che per tanto tempo sono state autoreferenziali, così come sta dimostrando anche la relazione del commissario di Bankitalia che ha certificato nel corso del tempo gli andamenti della malagestione della banca. Penso che noi dovremmo avere una grande responsabilità, perché riconoscere

dei cittadini e di un rapporto tra banche e territorio, che deve tornare ad essere positivo perché i territori hanno bisogno di una politica finanziaria che che li possa sostenere. Se, invece, c'è chi sceglie ancora, per il gusto della polemica e per qualche voto in più, di fare puramente polemica senza riconoscere un passaggio così importante, vuol dire che non ha a cuore l'interesse dei cittadini, ma solo l'elemento di speculazione politica. Questo porterà poco lontano e sicuramente

a verificare se, all'esito dell'approvazione del decreto e dell'ulteriore conversione in legge, ci sarà un'ulteriore sperequazione da parte del sistema il mio intervento si concentra Non entro nel merito di tutte le questioni tecniche e giuridiche che riguardano le novità introdotte dal decreto

per quanto riguarda le banche, dei passaggi di tutela giurisdizionale. Questo per noi è incostituzionale e, per questo, abbiamo votato a favore delle questioni pregiudiziali proposte anche dagli altri Gruppi d'opposizione.

che hanno anche loro il diritto di soddisfare i propri crediti in maniera efficiente, così come con questo decreto si ritiene di poter fare solo per le banche. Pensiamo a quanto sia frustrante, in un momento di crisi economica come quello attuale, per le imprese riscuotere i propri crediti. Faccio solo l'esempio dei crediti verso le pubbliche amministrazioni: un'impresa creditrice verso le pubbliche amministrazioni si trova di fronte ad una serie di ostacoli notevoli. Penso al sistema dei debiti degli enti locali e territoriali: molto spesso ci si trova di fronte all'impignorabilità di somme, molte altre volte ci si trova di fronte

quotidianamente per garantire lavoro, sviluppo e crescita economica. In questa direzione, con questa *ratio*, vanno letti alcuni emendamenti che,

a emendamenti come il 4.15, che introduceva un riparto, anche parziale, delle somme realizzate nell'ambito di procedure esecutive, anche in pendenza di controversie tra creditori concorrenti o tra creditori e debitori; crediti non totalmente contestati, ma solo parzialmente, di poter dare una accelerazione e garantire una riscossione, anche parziale, nei confronti dei creditori che questo diritto vedono compresso con il sistema attuale. Ricordo poi gli emendamenti, sempre all'articolo 4, con i quali si è cercato di accorciare notevolmente i tempi delle procedure esecutive immobiliari. È vero che negli ultimi anni ci sono stati una accelerazione e un miglioramento in termini di tempistica rispetto alle vecchie procedure esecutive, che duravano oltre dieci anni e che, invece,

di accelerare i tempi del processo esecutivo immobiliare, non solo facendo dei salti tesi alla degiurisdizionalizzazione a favore delle banche, ma anche cercando di snellire ulteriormente le procedure esecutive, addirittura potendo evitare una serie di rinvii da una udienza all'altra e cercando di partire da subito con l'iscrizione a ruolo,

attutire la logica della svendita degli immobili, cercando di valorizzarli il più possibile. E ricordo che gli immobili oggetto di procedure esecutive immobiliari

sulla base di questa funzione, che deve essere riconosciuta sì agli istituti di credito, ma anche agli imprenditori, che sono la linfa vitale della nostra economia, e soprattutto alle piccole e medie imprese. la Commissione prima, con passaggi farraginosi e certamente frustranti per chi si era posto l'obiettivo di migliorare il testo, e poi addirittura il voto di fiducia sul maxiemendamento che sta per arrivare, annullano

dai cittadini e dagli utenti dello stesso mondo bancario, contigui ai consigli di amministrazione dei diversi istituti di credito e insensibili ai drammi di soci e correntisti. E si rileva questa distanza anche dinanzi proposte emendative costruttive e non ideologiche che ho illustrato prima. Si voleva solo sveltire il processo esecutivo e aiutare gli imprenditori in crisi, ma non si è voluto prestare ascolto a questo tipo di istanze. Quindi, potremmo concludere che quel solco che segnava la distanza tra Governo e cittadini è diventato prima una trincea e oggi un vero e proprio fossato e i risultati del 5 giugno sembrano attestarlo plasticamente. PRESIDENTE. MPL))*. Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, vorrei fare una breve retrospettiva. Ricordo quando di questa vicenda si è iniziato a parlare: eravamo alle porte della pausa natalizia e siamo tutti stati immersi in complicatissime questioni riguardanti il diritto bancario italiano ed europeo. All'inizio è stato fin troppo facile puntare il dito contro l'Europa e dare agli euro-burocrati la colpa di quanto avvenuto a Banca delle Marche, Carichieti, Carife e Banca Etruria. Già allora però si ponevano alcuni quesiti che non hanno fin qui avuto risposta: se il Governo Renzi era così contrario alle norme europee sul *bail

Perché non ha usato la forza della sua rappresentanza in seno alle istituzioni comunitarie, come invece ha fatto o almeno cercato di fare E ancora, colleghi, una volta che queste regole, nel bene o nel male, sono state emanate, perché nel trasferirle nell'ordinamento italiano si è andati avanti a due velocità, a seconda che si trattasse di amministratori o di risparmiatori? Come abbiamo cercato di ricordare invano al Governo in quei giorni, le due direttive gemelle, una sulle procedure di risanamento delle banche, l'altra sulla garanzia dei depositi dei risparmiatori, erano state approvate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea non a caso - in contemporanea, lo stesso giorno. Senza l'una, l'altra sarebbe stata non solo inutile, ma dannosa. Lo si è visto dopo pochi giorni con quello che è successo nel nostro Paese. Il Governo infatti, per una fortuita casualità, si è ricordato di recepire frettolosamente la direttiva sul risanamento delle banche (il 16 novembre 2015), appena in tempo per applicarla ai casi delle quattro banche in oggetto e, in particolare, di Banca Etruria (il 22 novembre 2015). Per un'altra fortuita casualità, invece, ha dimenticato nei cassetti di Palazzo Chigi, fino all'8 marzo 2016, la direttiva che creava il sistema di garanzia dei depositi dei risparmiatori, quali, infatti, si sono visti azzerare i risparmi dalla sera alla mattina. Anche qui, però, serve un po' di precisione nella ricostruzione. Non tutti i risparmiatori si sono visti azzerare i risparmi, perché dalle notizie che sono trapelate sulla stampa (le avete lette tutti) dalla procura di Arezzo si sospetta che alcuni risparmiatori eletti siano stati avvisati per tempo di ciò che sarebbe successo. La presunta soffiata avrebbe sottratto alla banca 288 milioni di euro in poche settimane, creando una voragine nei conti e accelerando ulteriormente il *default* dell'istituto toscano. Il tutto a dispetto degli ignari che a quelle banche avevano affidato i risparmi di una vita. A seguito del "fallimento guidato" di Banca Etruria & Co.

a partire dalla scorsa legge di stabilità si sono susseguite rassicurazioni su una imminente soluzione; dall'altro, si è più volte lasciato intendere che questi risparmiatori fossero colpevoli di di «un investimento sbagliato». Alcuni membri del Governo li hanno addirittura paragonati a degli «imprenditori che si assumono il rischio di impresa». Sarebbe facile ironizzare sulla riscoperta, d'un tratto, delle regole del mercato liberale. Noi, che forse abbiamo qualche titolo in più per parlare di leggi del mercato e sostenere che esse sono uguali per tutti e che chi più guadagna più rischia, diciamo con chiarezza che queste regole sarebbero valse qualora i risparmiatori aretini fossero stati consapevoli di ciò che stavano sottoscrivendo. Da quanto emerge dalle indagini e propagato dalla stampa, in questo caso le cose sono andate in modo piuttosto diverso. I dirigenti di Banca Etruria avrebbero portato al fallimento l'istituto finanziario a suon di concessione di lauti finanziamenti a imprese alle quali, poi, chiedevano in cambio false consulenze. dirigenti avrebbero sollecitato i sottoposti affinché vendessero le obbligazioni subordinate allo sportello. I funzionari, poi, pur di ottemperare all'ordine, avrebbero addirittura falsificato i profili di rischio dei clienti, attribuendo loro lauree e titoli di studio mai conseguiti. Sono stati ritrovati documenti in cui pensionati di novantatré anni dichiaravano, a loro insaputa, di non voler ritirare i soldi investiti per i dieci anni successivi. Evidentemente, la loro aspirazione di vita è abbastanza lunga e ciò mi ricorda quello scrittore tedesco che diceva che a cento anni non si preoccupava di morire perché leggeva i necrologi e scopriva che alla sua età non sono poi tanti quelli che muoiono. Elementi come questi non possono che testimoniare una pesante responsabilità da parte dei vertici di Banca Etruria. Davanti a questo genere di "fango" riportato dai giornali (così è stato definito dal Presidente del Consiglio in quest'Aula), lo stesso *Premier* ha pensato, in principio, di scaricare ancora una volta la patata bollente sull'onnipresente Raffaele Cantone, una sorta di *passepartout*: a lui il noioso e ingrato compito di operare la selezione tra i risparmiatori che - cito - rientravano nella categoria

Colleghi, la percentuale di clienti presumibilmente truffati da Banca Etruria sembra essere talmente alta che persino i nuovi vertici della cosiddetta *good bank* hanno tentato invano di accelerare i tempi, proponendo al Governo di provvedere a un primo parziale rimborso finanziato con risorse autonome. Man mano che le indagini procedevano e le relazioni della Banca d'Italia venivano rese note, anche il Governo ha dovuto prendere atto dell'insostenibilità di questa vicenda, tanto da mettere da parte Cantone, dare il benservito all'ambasciatore Sannino (allora capo della Rappresentanza italiana presso l'Unione europea definito troppo morbido nelle trattative con l'Europa) e trasformare magicamente un tecnico governativo di alto livello come Carlo Calenda in diplomatico della Repubblica. A Carlo Calenda - lo abbiamo capito in seguito - l'ardua missione di fare la voce grossa in Europa per ottenere maggiori risorse evitando di incappare nell'ostacolo degli aiuti di Stato. Soldi, questi, destinati al risarcimento degli «scellerati investitori di Banca Etruria». I 100 milioni stanziati in sede di legge di stabilità - lo avevamo detto in tempi non sospetti credo che il presidente Sangalli mi può essere testimone - sarebbero stati assolutamente inadeguati a ripianare un buco di 328 milioni di euro. A tanto ammontano le perdite subite dai risparmiatori. Non a caso, colleghi, la nomina dell'attuale ministro dello sviluppo economico Calenda nella prestigiosa Rappresentanza di Bruxelles risale al 19 gennaio, il nulla osta dell'Unione all'aumento di capitale a 300 milioni di euro del Fondo destinato ai risparmiatori è arrivato il 20 aprile, e Carlo Calenda ha restituito la feluca solo 16 solo 16 giorni dopo per essere promosso a capo del Dicastero di Via Veneto. Il 29 aprile, giunti oramai alla ventiduesima «settimana decisiva» - perché ogni settimana era annunciata il decreto per gli indennizzi ha finalmente visto la luce. Meglio tardi che mai, avranno pensato i 10.559 correntisti protagonisti di questa amara vicenda. Certo, perché non sapevano ancora che nemmeno questa sarebbe stata la volta buona - cerco di parlare con linguaggio comprensibile al Governo - e che si sarebbero trovati davanti a numerosi bivi, molti dei quali li avrebbero portati in strade senza uscita. portati in strade senza uscita. Ad esempio, tra coloro che avevano effettuato l'investimento prima del 12 giugno 2014 e coloro che lo avevano sottoscritto dopo si fa una grande differenza. La data spartiacque - non a caso - è quella in cui sono state pubblicate sulla *Gazzetta* dell'Unione europea le due direttive gemelle. La seconda categoria potrà accedere solo alla lunga e farraginosa strada dell'arbitrato, mentre per chi ha investimenti precedenti al giugno 2014 si apre anche la strada del risarcimento automatico. Automatico sì, ma con molti se: se il reddito è inferiore ai 35.000 euro; se il patrimonio mobiliare è inferiore ai 100.000 euro; e in ogni caso, nella più rosea delle ipotesi, il rimborso non potrà essere maggiore dell'80 per cento di quanto investito; al netto di oneri e spese di acquisto; al netto della differenza fra il rendimento complessivo dei titoli incriminati e il rendimento dei titoli di Stato. E se mai capitasse che questa differenza fosse a vantaggio dell'investitore, questa verrà decurtata dalla somma risarcita. A chi opti per una delle due soluzioni, poi, verrà automaticamente preclusa l'altra. In sostanza, traducendo in italiano - e chiedo al Governo

ma in fondo se guadagnate più di 1.500 euro al mese o avete altri investimenti finanziari del valore di un *box* auto a Roma, oppure se quando siete stati ingannati dalla vostra banca non eravate coscienti che era entrata in vigore una direttiva europea, che il Governo non avrebbe ratificato se non quando utile per il caso Etruria, allora, la vostra truffa è nulla e voi non avete bisogno di essere risarciti». Verrebbe da commentare: «Non è questo il mercato, bellezza!». Colleghi, con questo sistema si disincentiva di fatto l'accesso all'arbitrato affabulando i risparmiatori con un sedicente rimborso automatico come ho cercato di dimostrare, automatico non è. Si prendono quindi due piccioni con una fava: si illudono i risparmiatori di poter recuperare almeno in parte quanto perso e si evita - come sarebbe avvenuto grazie agli arbitrati - di rendere nota la percentuale degli investitori spericolati, come definiti dal *Premier*, e quindi si evita, per differenza, di sapere quanti sono gli investitori truffati da Banca Etruria. A questo punto ci siamo illusi di poter esercitare il nostro ruolo di legislatori, modificando il decreto durante l'esame in questo ramo del Parlamento, ma anche l'ultima fiammella di speranza si è spenta quando abbiamo compreso che ogni ipotetica modifica doveva rientrare in emendamenti sottoscritti dai relatori, previo nulla osta del Governo. Arrivati in quest'Aula, con metodo altrettanto democratico, si annunzia l'apposizione della questione di fiducia in entrambe le Camere. Colleghi senatori, rappresentanti del Governo, dopo questa estenuante vicenda, di cui ancora molto si dovrebbe conoscere e molto si dovrebbe discutere, non riesco proprio a trovare alcuna motivazione ragionevole per votare a favore di questo provvedimento. Per me che faccio parte dell'opposizione è scontato, ma forse anche qualche collega della maggioranza ci dovrebbe pensare. In questo caso, concedere la fiducia in bianco all'Esecutivo non è soltanto un errore, è davvero qualcosa di più. E forse varrebbe la pena non avere correlazioni di carattere "morale" con un provvedimento di questo tipo. *(Applausi dal sarebbe stato interessante che i parlamentari del PD, così bravi a difendere questo provvedimento, fossero venuti ieri mattina fuori da questo palazzo, dove c'erano gli investitori che sono stati platealmente truffati e ora anche ignorati,

bene? Loro vanno in televisione e dicono che quei risparmiatori si sono comportati da speculatori, hanno voluto guadagnare di più e allora hanno accettato anche il rischio. Sarebbe stato interessante, invece, avere qui il caro

E bisognerebbe chiedere delle spiegazioni su come mai gli amministratori, più cinque sindaci, tra i quali c'era anche il padre della Boschi (persona per bene), si sono concessi 198 posizioni di fido per 185 milioni di euro. Ne hanno utilizzati 142 e 108 non sono tornati indietro. E allora perché non torna indietro ai nostri poveri concittadini

con la complicità del Governo e con il padre della ministra Boschi, persona perbene, che sedeva in quel consiglio di amministrazione da anni, e non negli ultimi sei mesi, avete truffato quelle persone

non si chiamano Marchionne né "Riva d'Ilva", allora tutto tace, tutto si infogna e si insabbia. Questo state facendo. Se non è così, richiamo con l'Adusbef tutti i risparmiatori. Abbiate il coraggio, la faccia e la trasparenza di portare Pierluigi Boschi, padre della Boschi e persona perbene, la Boschi stessa, Padoan, Renzi e tutta la maggioranza fuori dai palazzi senza scorta, per andare a parlare con quella gente a cui state rubando ancora i soldi. Siete disonesti e in quest'Aula, nei programmi televisivi e sui giornali non riuscite ad abbracciare l'onestà, neanche di fronte alla più plateale evidenza dei fatti.

io, così come tutto il Gruppo di Forza Italia, non condivido il provvedimento in esame e cercherò di spiegare i motivi. credo sia giusto dare atto innanzitutto ai relatori Zeller e Mauro Maria Marino - e quest'ultimo anche nella sua veste di Presidente della Commissione - e al sottosegretario Baretta che in Commissione è stato consentito all'opposizione di lavorare sul provvedimento e di esprimere le sue opinioni, opinioni che talvolta sono state tenute in considerazione - secondo noi, troppo poco

Mi auguro - e conto sulla correttezza del presidente Marino, del suo correlatore Zeller e del sottosegretario Baretta - che il maxiemendamento che arriverà tra poco al nostro esame tenga conto realmente del lavoro compiuto e degli emendamenti che in Commissione sono stati approvati. Passiamo al provvedimento. La prima parte del provvedimento, sostanzialmente, attraverso una serie di articoli, tende a supplire a una delle grandi carenze del nostro Paese, e cioè il fatto che, quando un creditore trova un debitore che non vuole o non può pagare, in realtà, per recuperare il proprio credito, i tempi sono biblici. La strada maestra sarebbe stata quella di fare una vera riforma della giustizia civile, sia nelle norme che nel funzionamento. è una risposta parziale a un problema che in realtà esiste. Qual è il problema che penso sia giusto sottolineare in questa vicenda? Quando una grande o una media impresa o un'impresa strutturata si confronta con la banca, che è in questo caso il creditore, è attrezzata: ha un avvocato, sa di cosa parla, ha un potere contrattuale Ma quando il debitore è un piccolissimo artigiano, un piccolo imprenditore che ha tre o quattro dipendenti,

emendamento non è stato approvato. Quello che chiediamo è che, al di là di alcuni miglioramenti che sono stati apportati (sono stati concessi tempi

Per quanto riguarda la questione dei rimborsi, si è cercato di lavorare perché i paletti, che - come il relatore Marino ha correttamente ricordato

i truffati più deboli, rispetto a quelli che magari sono di più. Vorrei sottolineare due aspetti sotto questo punto di vista, che sono molto importanti. In primo come ha ricordato il relatore, è indispensabile che l'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione sia effettivamente realizzato dal Governo e che quest'ultimo faccia in fretta

La Commissione finanze ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che dice che non devono essere tassati. Mi auguro che venga tenuto in considerazione questo aspetto. Vorrei poi passare a un altro punto che mi sembra rilevante, l'articolo 12, sul quale anche il relatore ha posto l'accento.

L'uso delle tecnologie moderne comporta delle ristrutturazioni, che comportano dei sacrifici per il numero delle persone che possono lavorare.

La seconda motivazione, che è ancora più rilevante, è che le persone

dal mercato se si licenziano i lavoratori e coloro i quali gestiscono le aziende, magari uno o due anni prima

dovrebbe dire che il settore bancario, dove saranno apportate grandi ristrutturazioni e dove ci sono persone che sono state molto bene negli anni scorsi, verrà da noi aiutato a ristrutturarsi e a migliorare, in modo da creare i minori danni sociali possibili.

ho ascoltato il dibattito e alcuni interventi mi hanno lasciato molto sorpreso. due minuti, perché credo siano state fatte valutazioni assolutamente non condivisibili e lontane dalla realtà. Desidero, però, in premessa dare atto al Governo, al presidente Marino e al relatore Zeller di aver consentito di svolgere in Commissione un lavoro molto proficuo, proficuo, che ha visto tutte le forze di maggioranza e di opposizione contribuire positivamente al lavoro e al miglioramento del provvedimento oggi in esame. atto al collega Carraro della sua correttezza, come sempre, perché interviene allo stesso modo in Commissione e in

assolutamente lontane dalla realtà, visto che il tema degli interventi sull'intero sistema del credito e sul rafforzamento del sistema bancario è teso a consentire il miglioramento del sostegno all'economia reale; dall'altra parte, i provvedimenti adottati, con la legge Sabatini e con il superammortamento, hanno determinato risultati molto positivi nel settore dei macchinari industriali, tanto che

con quella degli altri Paesi europei e negli ultimi venti anni registriamo una situazione di palude, di ristagno, che è un problema vero. Probabilmente ha ragione chi tra gli osservatori ha individuato la causa vera nel blocco, nella paralisi, nella mancanza di riforme che alla che alla fine, nella competizione con la globalizzazione, e quindi con una competizione globale, tutto il nostro sistema Paese con le sue arretratezze (dalla pubblica amministrazione, al mercato del lavoro, alla formazione, al fisco e a quant'altro) ha scontato e continua a scontare. E solo adesso con la vigorosa stagione di riforme stiamo cercando di uscire da questa difficoltà. Sul tema del risparmio vorrei che, in una fase iniziale, abbiamo avuto una ricomposizione dello *stock* del risparmio delle famiglie che lo avevano consumato negli anni della crisi. In realtà i dati ci dicono che la ripresa del PIL, proprio a fronte delle difficoltà del commercio globale, è sostenuta dalla domanda interna, dalla ripresa dei mutui edilizi, del credito al consumo, dall'acquisto di automobili, di case e così via. C'è, in realtà, una ripresa di fiducia e di spesa, favorita anche da alcuni provvedimenti. È vero - come lei stesso ha sottolineato - che una parte importante

al sostegno ai redditi medio-bassi, al rinnovo dei contratti che, in realtà, servono non solo a dare spinta economica al Paese e fiducia alle persone, ma anche e soprattutto hanno la valenza di provvedimenti di giustizia sociale non più rinviabili. che oggi ci accingiamo a convertire in legge è un provvedimento importante che si colloca all'interno di un complessivo percorso di riforma del settore creditizio italiano, che a sua volta si inserisce nel più ampio processo in atto a livello europeo. A partire dagli inizi del 2015, il Governo ha avviato un processo di riforma teso a rendere gli istituiti creditizi più competitivi e a potenziarne il ruolo di supporto all'economia reale. In particolare, vanno ricordate la riforma delle banche popolari e la più recente riforma delle banche di credito cooperativo. Gli effetti positivi dell'azione riformatrice messa in campo con questi provvedimenti si osserveranno nei prossimi mesi, contribuendo in modo deciso al rafforzamento di tali banche e, in generale, del sistema bancario italiano, promuovendone il consolidamento patrimoniale, il miglioramento dei modelli di *governance* e dei sistemi di valutazione del merito di credito delle imprese, nonché l'aumento dell'offerta di finanziamenti. All'interno di questa strategia è bene ricordare che il Governo è poi intervenuto con diverse misure sul principale ostacolo alla ripartenza del credito, rappresentato dalla mole dei crediti deteriorati accumulatasi nei bilanci delle banche. In proposito, voglio ricordare il decreto-legge n. 83 del 2015 (cosiddetto decreto fallimento), che ha introdotto misure per rendere più efficienti il recupero dei crediti e facilitare il ricorso a forme negoziali di risoluzione delle crisi d'impresa, prevedendo la deducibilità piena e immediata delle perdite su crediti. Con quest'ultima previsione il trattamento fiscale delle svalutazioni sui crediti è stato allineato a quello degli altri principali Paesi, consentendo di accrescere gli accantonamenti sui prestiti deteriorati e di ridurre i disincentivi alla loro cessione. Il successivo decreto-legge n. 16 del 2016 (cosiddetto decreto banche) ha previsto un meccanismo di garanzia dello Stato, a prezzi di mercato, a copertura delle *tranche senior* emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, realizzate a fronte della cessione da parte di intermediari finanziari di portafogli di crediti in sofferenza: un ruolo centrale nel favorire la cessione dei crediti non performanti e la creazione di un mercato efficiente di tali crediti, che potrà avvenire grazie all'importante ruolo che sarà chiamato a svolgere il Fondo Atlante. Si tratta di una strategia di ampio respiro che, in linea con le nuove misure europee, dovrebbe ricostruire un nuovo rapporto tra investitori e settore creditizio e tra quest'ultimo e l'economia reale, in modo da allinearli alle esigenze dell'attuale congiuntura economica. Una positiva notazione sistemica riguarda infine la circostanza che il provvedimento in conversione si inserisce in un complessivo ripensamento culturale delle diverse procedure che si attivano a fronte dei mancati pagamenti dei crediti. Il decreto-legge, infatti, arriva a poca distanza di tempo dal disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza dove, in linea con l'orientamento adottato dai principali ordinamenti europei, si è tentato di esprimere una nuova visione dello stato di difficoltà finanziaria, anche grave, visto come una possibile evoluzione fisiologica del ciclo dell'attività aziendale, da prevenire o gestire al meglio. Nel merito delle singole disposizioni, sono importanti le misure sulle procedure di insolvenza e sulle procedure esecutive, che si aggiungono a quelle già varate alcuni mesi fa, che, insieme all'istituto del cosiddetto patto marciano, contribuiranno a semplificare gli adempimenti e a snellire le procedure per il recupero dei crediti. Il complesso degli interventi avrà ripercussioni positive sull'economia reale in quanto le banche che rientrano più facilmente dei loro crediti avranno a disposizione spazi maggiori in bilancio per erogare prestiti alle imprese. Per quanto riguarda le ricadute sul sistema produttivo, vorrei ricordare un dato. La situazione italiana relativa ai crediti in sofferenza presenta delle peculiarità rispetto agli altri Paesi. Una risposta coerente non può che muoversi lungo due direttrici: velocizzare il recupero dei crediti delle banche verso le imprese, allineando i tempi italiani alle richiamate *best practice* internazionali; rendere più flessibile il sistema delle garanzie che assistono i finanziamenti, in modo da facilitarne l'ottenimento da parte delle imprese. La normativa introdotta e oggi in discussione è costruita intorno a queste due direttrici, rispondendo così a un'esigenza più volte rappresentata dalla classe imprenditoriale, cioè restituire efficienza e redditività al sistema creditizio in modo da garantire maggiore disponibilità di credito e migliori condizioni, a beneficio dell'economia reale. In particolare, le misure adottate potranno avere un impatto positivo non solo sull'apertura di nuove linee di finanziamento, ma anche per la rinegoziazione dei finanziamenti in essere. Grazie al testo in esame, sarà più facile per le imprese ottenere finanziamenti dagli istituti di credito, che possono contare su procedure semplificate e celeri per recuperare le somme erogate in caso di inadempimento nel pagamento delle rate. Il patto marciano prevede l'assegnazione stragiudiziale degli immobili dati a garanzia di un finanziamento ed è la novità più rilevante tra quelle del decreto-legge. prevede la possibilità che, a fronte di un finanziamento, le parti stipulino un contratto di cessione di un bene quale garanzia della restituzione. In caso di inadempimento del debitore, la banca entra in possesso del bene con una procedura molto semplice, senza il passaggio per il sistema giudiziario; al debitore spetta comunque la differenza tra debito residuo e il valore del bene, bene, che viene stimato da un perito indipendente, nominato dal giudice. Per il poco tempo a disposizione non mi dilungherò su altri aspetti importanti, che però sono stati sottolineati da vari interventi dei colleghi e dei relatori. Importanti sono, ad esempio, le misure che hanno impatto sui contratti di finanziamento già stipulati e sulla rinegoziazione di questi contratti; le misure di modifica della legge fallimentare e le procedure concorsuali, così come l'impatto che hanno altre misure importanti come il pegno non possessorio. Nella sostanza, il provvedimento in esame introduce elementi di riequilibrio funzionali del sistema giuridico ed economico in grado di favorire un effettivo fattore di sostegno all'economia reale, contribuendo al rilancio del tessuto produttivo del Paese. Si bilanciano gli interessi in gioco salvaguardando i principi di buona fede e correttezza contrattuale. Nell'attuale contesto economico è determinante assicurare che, a fronte di una corsia accelerata per il recupero dei crediti, si introducano presidi in grado di generare benefici concreti per le imprese in termini di ammontare, costo e durata dei finanziamenti, che dovranno risultare maggiormente sostenibili per le stesse contribuendo, in coerenza con la linea adottata dalla BCE, a delineare una politica nazionale per il credito anticiclica.

credo che le perplessità espresse da più parti, soprattutto dalle forze di opposizione, in ordine a questo decreto-legge non siano fondate. Ritengo invece che che i nuovi strumenti introdotti con il decreto-legge e perfezionati dal nostro lavoro in Commissione porteranno l'Italia Non dobbiamo infatti dimenticare che da parecchi anni, se non decenni, sia in dottrina ma anche

urgerebbe anche un intervento complessivo in materia senza ricorrere allo strumento del decreto-legge, ma questo avverrà con la legge delega, che è in fase di preparazione, sulla riforma

perché anche in altri Paesi si cerca da anni di riformare il sistema delle garanzie senza però che finora i risultati siano stati molto lusinghieri.

Sia l'istituto del pegno non possessorio che la previsione del patto marciano rispondono a questa esigenza.

emendamenti della sua parte politica, la richiesta di prevedere in norma un obbligo per una parte contrattuale di concedere un trattamento di maggiore favore ad un debitore

nessun debitore accetterà un patto marciano se non avrà in cambio qualcosa di positivo come una dilazione della restituzione delle rate da parte delle banche, un miglior tasso di interesse o qualche altra contropartita. Se non è così, nessun imprenditore sarà così poco accorto da dare in garanzia un immobile

dannoso, perché avrebbe aperto a delle possibilità per i creditori inadempienti. Tutti sappiamo che il grande male in Italia sono non solo i tanti avvocati, dei quali uno il relatore, ma anche le tante possibilità che noi legislatori abbiamo introdotto negli ultimi decenni

instaurando procedimenti lunghi e costosi. Penso che la competitività dell'Italia soffra anche per questo motivo, perché non scriviamo le leggi in modo chiaro, inseriamo la possibilità di fare eccezioni dappertutto e rendiamo illeggibili i testi di legge. Con questo provvedimento, che tratta già una materia molto complessa, abbiamo cercato di semplificare al massimo possibile proprio per cambiare il modo di legiferare. Lo scopo del provvedimento non è solo la semplificazione, ma anche l'accelerazione. E si può accelerare unicamente se non vi è la possibilità di bloccare un procedimento da parte di un debitore.

abbiamo studiato e discusso a lungo una procedura che consentisse al debitore di bloccare il decreto ingiuntivo, offrendo, di iniziativa sua, un patto marciano, e costringendo in questo modo la banca a esprimersi sull'accettazione o meno di questa garanzia. Era un articolato lungo e complesso e, alla fine, insieme al Governo abbiamo deciso di abbandonare questa strada, per il semplice motivo

saremmo andati contro la finalità principale di questo decreto-legge: quella di facilitare, semplificare e accelerare. In questo senso abbiamo abbandonato questa strada, ma

coerenza. Con il sistema delle stime e con il rafforzamento delle garanzie di terzietà del perito abbiamo migliorato il testo evitando anche delle distorsioni. Una questione è rimasta incompleta.

non può trasferirsi l'immobile del debitore e, al contempo, fare l'intermediatore e il mediatore immobiliare.

sulla concorrenza o in un altro apposito provvedimento, perché il tema è stato ben posto dai colleghi dell'opposizione, e sicuramente va trovata una

Non è stato possibile perché il decreto‑legge non è la sede idonea per disciplinare un istituto così

a quegli interventi che ho ritenuto degni di considerazione, perché in alcuni casi ‑ mi dispiace dirlo ‑ mi sono trovato più di fronte a un comizio che ad osservazioni precise e puntuali.

E quando si dice che si è di fronte a degli interventi *spot* - permettetemi, con tutto il rispetto necessario - non si ha presente il quadro delle cose che stiamo facendo. Avevo utilizzato la metafora della perla la serie di provvedimenti danno veramente il senso di una visione d'insieme: soltanto per ricordarli,

con gli aspetti collegati della garanzia delle cartolarizzazioni e delle sofferenze. Per fortuna ci siamo trovati preparati su questi temi, perché

Infatti nella visione d'insieme si ha la capacità di cercare non di risolvere il singolo problema, pur degno di nota (come ha giustamente evidenziato nel suo intervento la senatrice che è quello che riguarda la specificità dell'area di Pizzoli), ma di intervenire in maniera sistematica a favore dei cittadini e dei risparmiatori. Tanto è vero che il grosso errore commesso dalla senatrice Blundo nel suo intervento è quando ha detto buona fede, perché ho visto che alcuni emendamenti sono stati presentati proprio perché c'era stata una cattiva interpretazione della norma, avendo chiaro dove volessero andare ma finendo coll'andare nel senso contrario).

ai 200 miliardi, di cui 83 netti), vi sia un abbattimento progressivo e velocissimo che porta a 165 miliardi se i tempi passano da sette a quattro anni. Questi sono gli elementi reali su cui ci dobbiamo concentrare e che hanno cercato di rappresentare l'elemento ispiratore dell'azione che i relatori, in accordo totale con il Governo, hanno effettuato. Rispondendo all'indicazione del presidente Carraro, vigileremo che ci sia una coincidenza tra il testo approvato in Commissione e il maxiemendamento, ma penso che ciò sia in linea con il comportamento

pubblico riconoscimento). Come detto all'inizio, siamo di fronte a una rivoluzione copernicana che riguarda il cambiamento del rapporto tra il cliente e le banche, come determinato dalla direttiva BRRD. Andiamo a gestire in via eccezionale una fase di transizione sapendo che l'eccezionalità non varrà più per il futuro, ma lo facciamo con coscienza di causa, convinti di dare un contributo significativo al sistema Paese, all'interno di un progetto complessivo di riforma bancaria e non come un singolo *spot*. Questa è la scommessa che ci stiamo giocando e penso che, continuando così, insieme la potremo vincere.

esprime parere di nulla osta rispetto ai profili di copertura con quattro osservazioni, che ci permettiamo di trasmettere al Governo perché ne tenga conto nel presentare alla fiducia dell'Assemblea il maxiemendamento. La prima osservazione riguarda

all'emendamento presentato dal Governo, la lettera *c)*. Alla lettera *c)*, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente comma 4», la parola: «valutazione» è sostituita con la seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa», sono sostituite con le seguenti: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore». Questa lettera è saltata nella trascrizione e noi lo facciamo rilevare al Governo perché eventualmente proponga

ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore, di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto». Per ragioni che hanno a che fare anche con profili di copertura finanziaria, noi proporremmo di tornare al testo valutato positivamente dalla 5a Commissione,

«Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto», mentre nel testo valutato dalla Commissione bilancio era scritto «Sino alla scadenza dell'ottavo mese successivo all'emanazione del decreto».

nota in calce alla relazione tecnica, verificata positivamente dal Ragioniere dello Stato e quindi bollinata. Il Ragioniere generale scrive quanto segue: «Si procede alla verifica positiva della relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo 12-*ter*, di cui si chiede lo stralcio per mancanza di copertura finanziaria, in quanto la cessione a banche e intermediari finanziari dei crediti d'imposta per interventi di riqualificazione energetica, essendo effettuata nei confronti di operatori finanziari e non dei fornitori, come previsto dalla richiamata norma della legge di stabilità 2016, determina, secondo le regole di contabilità nazionale, la registrazione di un prestito del soggetto finanziatore allo Stato per l'importo della cessione e un corrispondente trasferimento del controvalore dallo Stato al privato. L'effetto di tale operazione è peggiorativo del debito e del deficit per l'intero importo del credito ceduto». La Commissione ha preso atto di questa

Signor Presidente, il Governo accoglie le proposte e le osservazioni relative alle correzioni o ad integrazioni:

1.58, in cui nulla si dice essendo stato presentato un testo difforme rispetto al testo del maxiemendamento. Quindi la relazione tecnica analizza esprime un parere rispetto a un testo che è diverso dal testo del maxiemendamento. Tutto ciò fermo restando, l'eliminazione o il recepimento di quelli che sono stati i riferimenti del Presidente della Commissione bilancio, che ha giustamente sottolineato le differenze tra una cosa e l'altra, determinano non la semplice eliminazione di punti, tipo lo stralcio dell'articolo comportano l'introduzione di parole, sensi e pesi economici diversi rispetto a quello che è il maxiemendamento. Quindi, se il Governo intende risottoporci un testo modificato, perché il testo è modificato da un punto di vista quantitativo e qualificativo, ben venga, però, se il soggetto titolato,

proporre le modifiche e mantenere la fiducia che è stata richiesta, e non il Sottosegretario, che non ha la delega per porre la questione di fiducia, né tantomeno può modificare il testo di un maxiemendamento su un decreto-legge.

su cui abbiamo anche espresso il nostro parere, come ha riferito il Presidente, ma questo naturalmente ci porta anche ad alcune considerazioni di carattere procedurale, procedurale, ossia che ci dovrebbe essere una maggiore possibilità di esame dei testi, dato quello che è accaduto, e non essere lasciato all'estemporanea capacità dei componenti della Commissione bilancio di intervenire su un testo che, peraltro, in sede di merito, non hanno avuto la possibilità di esaminare definitivamente. Mi rivolgo anche alla Presidenza, perché valuti l'opportunità, la prossima volta, che ci siano tempi più congrui, e anche un giudizio da parte della Commissione di merito rispetto all'allineamento tra il testo approvato in Commissione perché è vero che il Governo può presentare quello che vuole, ma quando il Governo viene a presentare un testo e ci dice che è uguale a quello approvato in Commissione, è chiaro che ci dovrebbe essere, a questo punto, anche da parte della Commissione di merito, un esame per verificare se è vero, perché purtroppo non è la prima volta che capita che questo Governo ci presenti delle differenze senza annunciarle.

Calderoli, faccio notare che quando il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia, come si evince del resoconto, ha parlato di un testo che recepisce le modificazioni proposte dalla Commissione, esattamente ciò di cui si è fatto promotore il Presidente della Commissione bilancio, rilevando tre errori materiali che rendevano il testo non conforme a quello approvato dalla Commissione. Quindi

Grazie

la Commissione bilancio ha rilevato che ciò non ha conseguenze di carattere finanziario e, quindi, manteniamo il testo votato in Commissione.

solo chi non ha proprietà immobiliari per un valore fino a 100.000 euro e ha un reddito lordo IRPEF non superiore ai 35.000 euro. Chiedo ai senatori di sinistra che sostengono questo Governo di sinistra se hanno fatto due conti:

letti? I fischi di oggi vi hanno fatto capire che l'economia non riparte. Credete che questo decreto d'urgenza (non vedo urgenza rispetto a questa cosa, naturalmente) aiuterà l'economia a ripartire?

da cui provengo. Nulla contro la grande impresa, naturalmente, ma per Renzi è importante andare con l'amministratore delegato di una grande azienda in America magari, ma non pensare ai piccoli e medi imprenditori. Non è importante pensare ai commercianti

e non serve dire «ho fatto l'arbitro», non serve buttare sempre tutto sul ridere. I problemi del Paese sono molto seri. Di questo decreto-legge si è già detto molto questa mattina; io ho ricordato due cose, le più semplici da intuire e da comprendere, e mi auguravo che le capiste e le comprendeste anche voi.

veramente a chi è stato eletto contro la sinistra e che non può condividere questa sinistra: vogliamo continuare a dare la fiducia? Io capisco che le divisioni del Partito Democratico - con il massimo rispetto - sono all'ordine del giorno sui giornali, in televisione e nelle discussioni quotidiane fuori da quest'Aula, ma continuare a dare la fiducia a un Governo che fa il male di questo Paese? Le elezioni della settimana scorsa ci hanno detto che gli italiani non ne possono più. La luna di miele, quella del 40 per cento delle elezioni europee, è finita da un pezzo; adesso non ci sono più gli applausi, ma i fischi delle assemblee generali; non ci sono più i voti del 40 per cento, ma i voti a tutte le altre forze di opposizione.

Devo concludere, signora Presidente, ho finito il tempo. Fuori, tra la gente, la fiducia è già sparita, è evaporata, è diventata evanescente, esattamente come è evanescente non solo il Presidente del Consiglio, ma anche questa squadra. se chi fa la squadra è evanescente, inadeguato e non all'altezza, metterà intorno a sé, tranne pochi, rarissimi casi, una squadra composta da giocatori evanescenti. Mi piacerebbe che i parlamentari, anche di maggioranza, delle forze che sostengono questo Governo

per segnalare che noi in Commissione avevamo proposto degli emendamenti e degli ordini del giorno. Visto che si è parlato di situazioni di crisi di queste banche, tant'è che vengono previsti dei processi espropriativi espropriativi e la possibilità addirittura di trasferimento di un immobile dato in garanzia a favore della banca, per agevolare il recupero del credito della banca o comunque una patrimonializzazione di quel credito,

Faccio riferimento a due tristissimi e drammatici casi verificatisi in Veneto. Uno riguarda la totale *mala gestio* della questione delle banche popolari, sia della Banca popolare di Vicenza che della Veneto Banca.

A seguito di quei disastrosi decreti, attraverso i quali è stato previsto l'obbligo della trasformazione delle banche popolari, obbligandole quindi alla quotazione, siamo arrivati ad un valore delle azioni

Ma cosa è successo nel frattempo? Pur sapendo che si andava incontro a questo disastro, dovuto alle conseguenze di un decreto-legge che è stato approvato qui, nonostante ciò, la Banca popolare di Vicenza ha fatto 43.000 nuovi soci dal 2013 al 2014, sapendo benissimo che andavano incontro ad una situazione di totale disastro. Arriviamo quindi ad oggi con un sistema nel quale questi risparmiatori non sono stati assolutamente ascoltati non hanno avuto nessun tipo di ristoro. Non solo vi sono aziende che hanno perso dei valori importanti, ma stiamo parlando di singoli cittadini che hanno perso tutti i loro risparmi, i risparmi di una vita, che potevano essere dell'ordine di qualche decina di migliaia di euro. Ma, fossero anche state poche migliaia di euro, se quello era tutto il risparmio di una vita, per quella persona una situazione del genere è un disastro. Ricordiamo che negli Stati Uniti reati quali l'aggiotaggio, le false comunicazioni, il falso in bilancio, l'estorsione e la truffa avrebbero portato a pene da trent'anni all'ergastolo, quando invece qui in Italia per questo tipo di sono previste delle pene lievissime, con ciò concedendo a chi gestisce questi istituti bancari di fare praticamente quello che vuole, tanto poi le conseguenze sono irrisorie. Quindi ci troviamo adesso con 119.000 azionisti, con

a fare la dichiarazione di voto a nome del Gruppo. A me preme sottolineare che questo è un piccolo passo in avanti verso le riforme e che il nostro è un Gruppo nato per fare in modo che questa fosse una legislatura di riforme e che non vi fosse il solito scioglimento, per avere un'altra e continuare ad avere i poli contrapposti, uno contro l'altro, a giocare a chi fa meno, cioè al tanto peggio tanto meglio. Noi riteniamo - e invitiamo il sottosegretario Baretta

Debbo dire che il presidente Renzi ha preso questi pochi fischi in sostanza dicendo: «Se avete il coraggio fischiatemi, ma io vada avanti con le riforme».

Qualcuno diceva che bisogna tornare alla politica con la «P» maiuscola. Riteniamo di essere un Gruppo parlamentare per le riforme e quindi un Gruppo con la «G» la «P» e la «R» maiuscole, perché questo è il nostro obbiettivo e cercheremo di portarlo avanti, anche a dispetto di chi vorrebbe

firme, il Governo va a casa. Fantastico: sarebbe bello se fossimo in Francia! Peccato che non ci siamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)**.* La seconda premessa è che, da quando sono in Senato, cerco di ascoltare tutti i discorsi che vengono fatti, a prescindere dalla loro qualità, perché penso sempre che ci sia la possibilità di imparare qualcosa.

euro. Se, putacaso, avessi optato per il risparmio amministrato e avessi 30 milioni di euro in quello strumento finanziario, i proventi del risparmio amministrato non andrebbero nella dichiarazione dei redditi e quindi figurerei con una dichiarazione dei redditi pari

Vedete: qua la storia non insegna mai nulla, perché questo fatto per la prima volta è stato evidente negli anni Ottanta in Giappone, quando le banche facevano esattamente quello che hanno fatto in Europa e in Italia, ovvero prestavano soldi un po' a tutti. prestavano con tanta più manica larga, quanti più erano i soldi che venivano richiesti. In Italia succede la stessa cosa: la maggior parte dei soldi che le banche prestano, li prestano a chi ne vuole tanti. Le banche fanno meno storie per darne tanti e più storie per darne pochi, e quando te ne danno pochi chiedono anche delle garanzie. Ebbene, sull'onda di quello che successe in Giappone, l'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokio arrivò quasi a 40.000 punti (per capirsi adesso gravita a 16.700). Questo è quanto è successo quella volta, perché poi è scoppiata la bolla immobiliare: i valori immobiliari erano stati sparati verso l'alto e dopo sono crollati. È successo di nuovo pochi anni fa negli Stati Uniti e lo schema è stato uguale e naturalmente è successo di nuovo adesso, perché c'è ancora un problema di bolla creditizia. Il punto è che non si riesce bene a capire quanti soldi le banche hanno dato a gente che non è in grado di restituirli, soprattutto considerando azioni come quelle della Banca Boschi, alias Banca popolare dell'Etruria e del Lazio «nuova» (perché adesso si chiama Nuova Banca Etruria). Sono banche che hanno dato prestiti così

tu sei sottocapitalizzato, io ti giro un immobile mio, diventa tuo e automaticamente il tuo patrimonio sale. Permettiamo alle banche di mettere le mani facilmente sui beni mobili e immobili delle imprese, dopo aver toccato naturalmente quelli dei privati (cioè

o materie prime, deprimendolo ulteriormente, facendo scendere i corsi immobiliari e il valore delle materie prime e svalutando ulteriormente il patrimonio immobiliare che le banche stesse hanno, quindi in ultima analisi fanno un danno questioni di economia di base e non sono difficili da comprendere. Questo è il motivo per cui i provvedimenti che avete messo in fila per aiutare le banche non funzionano. Il vero motivo per cui tutto non funziona è che le banche stanno facendo la cosa sbagliata, cioè usano i tuoi soldi per fare profitto:

Una volta che ci siamo inventati di prendere a prestito il denaro dal futuro (chiamasi erogazione di mutui e prestiti), non possiamo più creare denaro; le banche non hanno mai avuto questo potere di creazione del denaro, però hanno il potere di distruggerlo.

quindi bisognerebbe limitare la possibilità delle banche di amministrare. Voi avete fatto esattamente il contrario: avete dato alle banche la possibilità di mettersi insieme perché diventassero più grosse nella speranza che chi aveva più soldi in pancia potesse aiutare chi ne aveva meno. aveva meno. Questo esperimento è stato già fatto nel Stati Uniti ai tempi della crisi immobiliare, quando hanno cercato di dare in pasto le ex sorelle (come Bear Sterns, Lehman Brothers, Merril Lynch, Morgan Stanley) a qualcuno di più grande. Infatti Bank of America ne ha preso un pezzo e Wells Fargo se ne è preso un altro. È andata a finire che Bank of America Wells Fargo non stanno andando bene, perché si sono prese il bubbone con tutto il suo carico di debiti. Vogliamo farlo anche qui? Ci state provando con le banche popolari. Avete cioè provato a mettere insieme (è bellissimo il matrimonio) la Banca popolare di Milano e la Banca popolare di Novara, che in realtà è fatta dalla popolare di Novara e da quella di Verona, San Geminiano e San Prospero, e da tutto quello che vi viene in mente. Il risultato di tutta questa bellissima operazione è che una volta le azioni di questo istituto valevano circa cento euro e adesso ne valgono

insieme. Queste cose sono state già dette non da me, ma da fior di analisti finanziari nel corso degli anni; quindi, continuare su questa strada significa continuare ad erodere il capitale. Sapete perché poi il bubbone è venuto fuori? Perché le banche sono state riempite di titoli di Stato grazie ai prestiti della BCE, dato che la BCE si è inventata che se si continua a battere moneta, finché qualcuno non si accorge che c'è una crisi di materie prime, e quindi non c'è inflazione, la si può creare dal nulla; quindi, le banche la prendono, comprano i titoli di Stato e speculano sul rendimento. Peccato che, da un lato, voi fate questo e, dall'altro, c'è l'esigenza di ridurre lo spread sui titoli di Stato. Quindi, si riduce il rendimento dei titoli; allora, se si dà da una parte e si strozza dall'altra, come minimo il risultato è zero. Anche questa non è molto difficile da comprendere; io non sono né un economista e neppure un analista finanziario, eppure queste cose le ho capite. Trovo altresì vergognoso che diate la colpa alla CONSOB. È vero, la colpa è anche sua, ma ce ne siamo accorti adesso che la CONSOB non vigila o vigila male? Al Governo ci siete voi e noi siamo all'opposizione - mi pare - quindi starebbe a voi fare in modo di rafforzare il potere di vigilanza di CONSOB e Banca d'Italia. Non è difficile.

e rinuncio ad un mio diritto». Avete trasformato il diritto di un risparmiatore di riavere quello che con fiducia ha dato alla banca, in un regalo. Trasformate un cittadino in un suddito. Questo non è un concetto difficile da comprendere,

Poi, però, non venite a lamentarvi se molte delle società, magari in accomandita semplice o Snc faranno la trasformazione in Srl per cercare di scaricare il loro rischio. Vogliamo fare anche questo? Questa si chiama distruzione del tessuto produttivo italiano. Eppure, con i piccoli non vi fate scrupolo mentre con gente come i Riva e l'ILVA vi fate tutti gli scrupoli di questo mondo. fronte ad un'azienda che perde 2,5 milioni al giorno, ancora trovate il modo di chiedere alle banche di fare prestiti ponte. ponte. Adesso si spiega perché voi volete così tanto aiutare le banche e perché le banche chiedono e ottengono. Se al sistema bancario si chiede di fare cose assurde come salvare

la ricapitalizzazione delle quote di Banca d'Italia, la ripulitura della quaterna delle banche, Montepaschi di Siena non si tocca e poi? Ci saranno altre banche ancora. A proposito, ma la vostra Commissione d'inchiesta sul sistema bancario il senatore Stefano Esposito, quello che ha detto che sarebbe stata fatta, incardinata e portata in Aula. Sì, l'ha detto, ma non ha detto quando. Infatti, stiamo ancora aspettando. Le persone perlomeno aspettano una cosa semplice: la verità. Bisogna avere il coraggio di dire ai cittadini che hanno perso soldi perché li hanno persi e non criminalizzarli dicendo che è un investimento di rischio. È vero, comprare un'obbligazione è un investimento di rischio, però lo si deve dire. Questo è il principio della trasparenza e dei moduli MiFID: io devo sapere esattamente dove mi stai facendo mettere i soldi. Quando questo viene meno, si parla di truffa, e un truffato va indennizzato al cento cosa che non è stata fatta. Però ditelo: «Noi siamo dalla parte del sistema bancario e chi se ne frega», così noi qui ci mettiamo tutti tranquilli e io non apro più bocca. Però non venite a raccontarci la favola, perché le favole qui non le vogliamo più sentire, ma soprattutto non vogliono sentirle le persone fuori di qui, perché ci sono migliaia di persone che hanno perso dei soldi e non vogliono sentirsi dire: «ti do la mancetta, basta che te ne stai buono». Questa è la cosa più importante che dovreste fare e spero ancora che la facciate. Grazie, dibattito sulla fiducia per qualche considerazione politica che potrà anche lasciare il tempo che trova, ma che, almeno per quanto riguarda, ritengo doverosa. Sul provvedimento hanno parlato altri colleghi che sono intervenuti. Ci sarà, immagino, una dichiarazione di voto di merito

facciamo una volta per uno, XVII).* Dicevamo che il Governo ha perso un po' la sua verginità su vicende bancarie e vicende petrolifere, che guarda caso sono le vicende classiche della politica: di

tutte le vicende del Monte dei Paschi di Siena, che sono altre, diverse e non risolte. Ricordo, ed è un po' un paradosso, che il presidente dell'Associazione bancaria italiana era Mussari. Lo ricordo nella scorsa legislatura veniva spesso nella sua veste istituzionale a colloquio con i Capigruppo per rappresentarci la preoccupazione della crisi bancaria; forse pensava alla crisi del Monte dei Paschi di Siena che conosceva, essendo anche presidente di questo istituto E mi fa un po' ridere, in tempi di antipolitica e di rottamazione della politica, che dopo Mussari ed altri alla presidenza dell'ABI è dovuto andare un galantuomo che prima era un politico, l'amico Patuelli, cui rivolgo un saluto dall'Aula del Senato. È un paradosso, in un'epoca in cui i politici fanno schifo e sono una casta, che il mondo bancario, dopo una crisi

d'Italia, adibita alla vigilanza se non ricordo male (vero, senatore Tremonti?). Siccome non aveva vigilato su quello che accadeva al Monte dei Paschi la fecero presidente della RAI. Adesso anche la Banca d'Italia avrebbe molte cose da spiegare: cosa ha fatto Visco? Cosa hanno fatto?

Peraltro la Banca d'Italia ha molto da farsi perdonare. Leggevo le notizie delle banche venete di Zonin, che rappresentano un altro scandalo bancario: ma avete letto quanti dirigenti della Banca d'Italia venivano assunti poi da Zonin? Ma che vergogna che vergogna questa Banca d'Italia! Che lerciume! Noi veniamo additati come politici perché siamo la casta delle caste e quelli della Banca d'Italia? Passavano dalla Banca d'Italia alle banche di Zonin. Ed erano quelli che dovevano controllare! Che Zonin abbia fatto delle cose non corrette mi auguro che sia la magistratura a sancirlo, ma alla Banca d'Italia chi glielo presenta il conto? Vergognati di questo passaggio da Banca d'Italia alle banche venete che hanno impoverito i cittadini, come sanno i colleghi veneti, ma lo sappiamo anche noi. Le azioni da 60 euro sono scese a 60 centesimi. La provincia di Vicenza e dintorni ha perso punti di PIL.

AL-A. Colleghi di AL-A, rendetevi conto di quello che vi dicono i signori del PD: dateci il voto al Senato, mai ai comizi non vi fate vedere perché se arriva qualcuno di AL-A a Napoli e a Cosenza non andiamo neanche al ballottaggio e a Cosenza vince addirittura il centrodestra al primo turno.

la confusione perché devi compensare, devi avere i voti e allora vai a inseguire l'uno o l'altro. Oggi serve. Non so se stasera sarà decisivo il voto di Tizio o di Caio. So che lo è stato, perfino per la leggina sulle Province del Friuli-Venezia Giulia.

E lo dico senza ritenere impresentabili quelli con i quali ho condiviso un percorso. Sono quelli che aiutate che vi tengono ai margini. Ho voluto fare una considerazione di natura politica. In fondo, questa sarebbe anche una Assemblea politica e democratica, oltre che un votificio su decretoni. Quanto alla discussione precedente: se il

nell'iniziare le dichiarazioni di voto al termine di una discussione generale che ha messo in evidenza molti aspetti, sia tecnici che politici,

che ha messo in evidenza il contesto politico nel quale questo decreto-leggeva a calarsi, è per me particolarmente impegnativo e serio. serio. Cosa non mette abbastanza in evidenza la discussione generale svoltasi finora? Che questo decreto-legge, sostanzialmente, non servirà a nulla. È costato tanta fatica a chi ha voluto produrlo, cioè al Governo, che però non si è preso la cura e la fatica di scriverlo correttamente e di affrontare il vero tema che

soprattutto alla Germania che, di fronte alla crisi e alle sofferenze bancarie nel proprio sistema del credito, ha risposto con l'unica misura seria che si poteva assumere: mettere risorse in quel sistema bancario per evitare la crisi sistemica, la crisi da paura e la crisi da incertezza.

vigilava poco o, almeno, vigilava con particolare attenzione su qualcuno ma molto meno su altri. Così è accaduto che un piccolo sistema di banche, quelle di quell'area territoriale che questa mattina descrivevo in discussione generale, tutte situate nel Centro Italia, tra la Toscana e dintorni,

collocato correttamente e difeso dall'azione delle leggi, dalla loro forza e da chi deve vigilare che quel risparmio venga garantito e difeso. Noi, invece, stiamo andando a legiferare, in virtù dell'iniziativa del Governo con il suo decreto-legge, su un sistema, quello bancario, che registriamo non essere stato opportunamente vigilato. Peraltro, Peraltro, abbiamo impedito al Parlamento di intervenire nel pieno di una crisi finanziaria come quella che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo

ha inoculato nel nostro sistema e nel risparmiatore. Come vedete, questo si sta ripercuotendo, anche per le omissioni di vigilanza di cui parlavo prima, su altri territori e su altri sistemi bancari, come come quello del Veneto, in capo alla Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca. Perché tutto questo? Perché la nostra risposta, a differenza di quella tedesca, opera su piccoli dettagli, che peraltro peraltro mandano in crisi, dal nostro punto di vista, quel sistema delle garanzie alle imprese a presunto vantaggio di un sistema di garanzie per il settore bancario

per consentire alle banche e al sistema economico di rivitalizzarsi. Giungo al dunque e alla parte conclusiva della mia dichiarazione di voto, che, come si può ben intendere, è nettamente contraria al

Attenzione che tra questi non c'è soltanto il sistema delle imprese, cioè un'impresa che fatica a recuperare il proprio credito da un'altra impresa, ma ci sono altri creditori, assai importanti, che sono i lavoratori, che nelle situazioni di prefallimento, di difficoltà e di crisi aziendale sono importantissimi. Noi a quei creditori non stiamo dedicando la stessa attenzione,

Tornando alla questione delle quattro banche e all'individuazione dei limiti patrimoniali e reddituali che danno diritto al rimborso forfettario, siamo sicuri che siano proprio giusti? Se una truffa c'è stata - e ci auguriamo che venga non solo stigmatizzata, come tutti facciamo, ma seriamente seriamente colpita - questa presunzione non può non estendersi anche nei confronti dei risparmiatori che non rientrano in quei limiti. Non è possibile, come dice il nostro presidente Marino, dire sempre che "il meglio è nemico del bene", perché questa volta il principio fondamentale di uguaglianza, messo così tanto in discussione, produrrà produrrà altri contenziosi che difficilmente potranno far dire a questo Governo che il decreto-legge in esame è servito alle banche, è servito a risolvere il problema dei risparmiatori truffati ed è servito al sistema economico, perché così non sarà. Noi abbiamo proposto l'eliminazione di quei limiti, ma mi rendo conto che il Governo questo poteva fare e questo ha fatto. il lavoro del sottosegretario Baretta, al quale riconosco non solo il merito di averlo seguito nel migliore dei modi, ma di essere uno dei pochi componenti del Governo ad avere la capacità di comprendere quanto questo decreto-leggesi riverserà

Ragioneria Generale dello Stato, che potevano in qualche misura agevolare una scrittura migliore e il perfezionamento di questo decreto-legge. E nessuno si nasconda dietro il fatto che le opposizioni si sono opposte, perché le opposizioni non hanno impedito al Governo di lavorare; anzi, hanno favorito la migliore delle soluzioni possibili per quei risparmiatori truffati e anche perché ci auguriamo che il provvedimento in esame possa davvero aiutare il nostro sistema bancario a risolvere i problemi.

che solo con un forte intervento di risorse economiche si può risolvere il problema. Il resto sono e saranno solo palliativi. Mi auguro che il Governo sia

il Governo e i relatori hanno sostenuto che il provvedimento in esame si colloca nel solco di altri interventi analoghi, promossi dalla maggioranza per sostenere la ripresa economica.

Secondo la vostra, le banche sono vittime delle imprese e degli artigiani che non pagano i debiti contratti e delle famiglie che non pagano puntualmente le rate dei mutui. Per voi i cittadini non sono vittime delle banche gestite in modo fallimentare e fraudolento, ma hanno perso i loro risparmi perché disattenti, impreparati e sprovveduti. Non è così:

Voi continuate a far ricadere il prezzo della crisi sui cittadini e favorite le banche nell'impossessarsi dei beni delle famiglie italiane in difficoltà. Infierite senza scrupoli su imprese, artigiani e famiglie che sono già in ginocchio approvate norme per rendere tali furti facili, veloci e legali. La crisi bancaria esiste non perché non si vogliono pagare i debiti contratti con le banche, ma perché non si è più in grado di farlo.

I cittadini italiani sono stretti nella morsa fisco italiano e banche e voi, con queste norme, la stringete ancora di più, probabilmente in modo irreparabile.

cassa, raccogliere denaro e affossare tutti noi, la nostra economia e le nostre famiglie. Signora Presidente, signori senatori, finora ho avuto difficoltà nel trovare ragioni per votare la fiducia a questo Governo e non ho trovato ragioni per votare la fiducia neppure in questo decreto-legge. Comunque cercherò di svolgere un intervento in qualche modo costruttivo.

perché è abbastanza evidente che quanto è in questo decreto-legge non basta e che quanto arriva da fuori sovrasta tutto in modo drammatico. Non è un mistero che entro luglio usciranno gli *stress* *test* europei, non è un mistero che il risultato sarà negativo per alcune banche europee ed è certo che sarà negativo per alcune banche italiane. Il fatto che la valutazione negativa sia anche fuori non è ragione per essere tranquilli, bensì lo è per essere preoccupati perché l'esperienza ci insegna che se la crisi è fuori viene aggravata e determinata proprio verso l'Italia. Si può dire che quei *test* hanno una base di metodo non corretta ed è vero, sono molto casuali. Dal primo *test* risultò tutto in ordine e tre mesi dopo fallì Dexia. Sono mentalmente sballati e tuttavia non si può fare un discorso di metodo per esorcizzarli e non credo che basti lo strumento denominato Atlante. Atlante è un accordo di cartello ma lo *stress* l'ha già subito, non è necessario lo *stress test* sulle banche italiane, è già stressato fortemente il signor Atlante.

Io ho l'impressione, e credo tutti l'abbiamo e anche voi l'avete, che la materia non sia stata gestita in questi lunghi mesi con la necessaria lucidità e con la necessaria capacità. Credo che non dobbiate e non possiate più limitarvi con gli *aut aut* di continui voti di fiducia. La materia esclude questa tecnica. La natura drammatica dei problemi esclude la sufficienza di questa tecnica d'Aula. Faccio una proposta: perché non vi aprite ad accettare anche le idee degli altri, le proposte degli altri? Ferme le divisioni politiche, tuttavia nella comune responsabilità verso le famiglie e il risparmio, perché non pensate davvero ad una Commissione interparlamentare che raccolga tutto quanto è necessario per affrontare una realtà che arriva e sarà molto più drammatica di quella che è stata finora? Resto dell'idea che le direttive europee non possano disapplicare la nostra Costituzione. Non credo che la direttiva sul risparmio possa, comunque, disapplicare l'articolo 47 della nostra Costituzione, l'articolo che definisce, come principio sacro, che la Repubblica tutela il risparmio.

Il decreto-legge al nostro esame è ovviamente diverso da quello licenziato solo qualche tempo fa, ma gli obiettivi sono identici: contribuire al rafforzamento patrimoniale degli intermediari finanziari, per ridurre, in qualche modo, l'impatto della crisi economica. Crisi in via di superamento, ma in modo talmente lento e tortuoso da non lasciare spazio al facile ottimismo. Del resto, le chiavi per risolverla con maggiore celerità non sono nelle nostre mani, né in quelle del Governo. Finché la politica europea sarà dominate dalle ossessive preoccupazioni tedesche, non sarà facile riconciliare politica monetaria e politica di bilancio, né individuare quell'ancoraggio - un *target* d'inflazione del 2 per cento - che dovrebbe essere il comune presidio per dare coerenza all'intero sistema. Purtroppo, almeno finora, si è verificato il contrario: da un lato una politica monetaria fin troppo espansiva; dall'altro una politica di bilancio tendenzialmente restrittiva, a livello globale. Ne è derivato un *surplus* delle partire correnti della bilancia dei pagamenti europei, che ha sostenuto il corso dell'euro nei confronti del dollaro, contribuendo ad inasprire la crisi dell'economia reale di tutta l'Eurozona. In un quadro così contraddittorio, il sistema bancario, non solo italiano, ha subito forti contraccolpi. Manca, infatti, una domanda di credito che sia, anche, solvibile, a causa del ristagno della domanda interna e delle difficoltà che molte aziende, poco internazionalizzate, incontrano sui mercati globali. Pesano inoltre i volumi dei crediti incagliati, che determinano fenomeni di spiazzamento patrimoniali, essendo necessario tenere immobilizzate riserve consistenti per far fronte al rischio che deriva da oltre 200 miliardi di crediti deteriorati, ai quali, nel periodo 2012-2015, si è fatto fronte con rettifiche di bilancio, che hanno compresso i relativi profitti, per un importo pari a 120 miliardi di euro. Quella residua esposizione, pari a circa 80 miliardi, quasi 5 punti di PIL, riduce notevolmente capacità di credito da parte delle stesse banche, costringendole alla ricerca di continue garanzie reali. La via maestra per risolvere un problema di questa natura sarebbe la riforma della giustizia civile, la cui lentezza è tale da aver fatto strame di ogni certezza del diritto. I tempi del processo sono talmente lunghi ed impervi da impedire qualsiasi soluzione delle relative controversie. Non è certo un caso se questo *handicap* costituisce uno dei principali ostacoli alla presenza di capitali esteri nel nostro Paese: non essendovi alcuna garanzia per la tutela dei singoli interessi, i grandi fondi d'investimento internazionali preferiscono rivolgersi altrove, confinando il nostro Paese in una sorta di limbo autarchico, che è la negazione stessa del principio di modernità al tempo della globalizzazione. Di fronte alle difficoltà di procedere lungo le linee di una riforma generale della giustizia civile, si è scelta la strada di un piccolo ritocco, che mira soprattutto ad accelerare le procedure per la riscossione di eventuali crediti. Si tratta di una procedura che ha una portata generale, come indicato dall'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame, ma la cui valenza più significativa è quella recata dal successivo articolo, che riguarda i rapporti tra il debitore e i singoli istituti di credito. Questo è infatti il rapporto prevalente che caratterizza l'economia italiana, piuttosto che quello relativo al singolo fornitore con il suo cliente. In questi casi lo strumento individuato è quello del pegno mobiliare non possessorio, vale a dire la costituzione di un pegno, a garanzia dei crediti o dei finanziamenti concessi, sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Beni che rimangono comunque nella disponibilità del debitore, costituendo l'oggetto dell'impresa. Pegno che si trasferisce automaticamente su oggetti della stessa specie e tipologia, ogni qual volta quelli originari sono utilizzati nel processo produttivo. L'istituzione del pegno determina un privilegio a favore del creditore, nell'eventualità in cui il debitore dovesse fallire. Il relativo credito è comunque iscritto nella massa passiva, ma in posizione diversa rispetto agli altri. l'eventuale escussione del pegno è rivolta solo a soddisfare le istanze di quest'ultimo. Poiché il nuovo istituto altera la *par condicio* dei creditori, è necessario che ad esso sia data adeguata pubblicità. Nell'articolo 3 è quindi descritta la relativa procedura. Se le garanzie per il creditore, che sono rappresentate dal patrimonio senza vincoli dell'imprenditore, si riducono, è bene che la cosa si sappia; che vi sia un regime di pubblicità adeguato al fine di tutelare i terzi in buona fede. In caso di inadempienza da parte del debitore, il creditore può procedere all'espropriazione forzata del bene pignorato. In questo caso, il pegno cessa di essere non possessorio e diventa possessorio, ma con le varianti proposte dall'articolo 2, riferite cioè al sistema di finanziamento da parte delle banche o altri istituti di credito. Da qui le motivazioni del precedente giudizio. Per consentire ai singoli istituti finanziari un maggior dinamismo gestionale, si stabilisce un nuovo canale di finanziamento, assistito da un sistema di garanzie più rapido ed efficiente. È utile aggiungere che simili disposizioni riducono l'esposizione al rischio di carattere sistemico e quindi dovrebbero - il condizionale è d'obbligo - contribuire al maggior rilancio degli investimenti, rendendo più agevole il finanziamento bancario. bancario. L'ultimo articolo recepisce alcune disposizioni comunitarie in tema di credito di imposta, prevedendone una diversa regolazione più in sintonia con le regole sugli aiuti di Stato. Dall'analisi delle singole disposizioni risulta pertanto evidente come il cuore del provvedimento sia rivolto essenzialmente ad alleviare il sistema bancario italiano, in un momento di particolare difficoltà, nella consapevolezza che solo un sistema bancario sgravato da costi indiretti possa contribuire con maggiore determinazione alla ripresa dell'economia nazionale. Nel condividere quest'interpretazione, non posso tuttavia non fare voti affinché lo stimolo che le singole banche possono esercitare su un'imprenditoria ancora troppo piccola si trasformi sempre più in una guida strategica. Abbiamo bisogno di avere banchieri sempre più amici delle imprese: più *tutor* che non semplici esattori. Nella speranza che anche questo provvedimento possa contribuire a questo più ampio orizzonte,

onorevoli colleghi, Sinistra Italiana voterà contro la fiducia al Governo e di questo certo non vi meravigliate.

in esame, perché il problema che poniamo e che abbiamo posto anche negli interventi in discussione generale è molto chiaro.

come uno degli strumenti che il Governo sta mettendo in campo per sostenere le piccole e medie imprese e aiutarle in un processo di ripresa economica, ma a nostro avviso le cose non stanno esattamente così

uomini e le donne, i lavoratori, gli artigiani e i piccoli imprenditori che, dalla mattina alla sera, non vedono

il trasferimento alla banca della proprietà di un bene immobile è alquanto penalizzante, perché noi immaginiamo facilmente le conseguenze per le imprese, in particolare per quelle piccole e medie che avranno ancor più difficoltà a rinegoziare i propri mutui.

della nostra platea di piccoli proprietari. Anche a questo riguardo sono state fatte delle piccole modifiche: da tre aste deserte si passa a quattro prima che il giudice possa

che tradisce l'operazione fatta, cioè quello che riguarda i risarcimenti alle migliaia di risparmiatori truffati dalle famose quattro banche. banche. A fronte di comportamenti illeciti a danno dei risparmiatori, sarebbe infatti stato doveroso da parte del Governo prevedere il rimborso integrale dei titoli, invece di fare cittadini di serie A e di serie B.

come un provvedimento di aiuto alle imprese, ai cittadini e per il risarcimento dei risparmiatori falliti, non tutela il risparmio, non aiuta e non garantisce i cittadini stessi

mi viene da sorridere quando in quest'Aula sento parlare di riforma della giustizia civile e penale da Gruppi parlamentari che al loro interno hanno dei rinviati a giudizio. Mi auguro che non ci mettiate

Tutti i provvedimenti che questo Governo ha fatto a favore delle banche non hanno portato assolutamente a incentivare il credito da parte delle banche alle imprese italiane. *(Applausi della delle stesse banche perché nei prossimi *stress test* le banche italiane saranno veramente in crisi. È di pochi giorni fa un articolo in cui si parla di rischio *bail in* per altre tre banche italiane: la Cassa di risparmio di San Miniato (che nel 2015 ha registrato un

In Italia abbiamo bisogno di altro, perché le banche che vogliono finanziare le imprese, lo fanno. Infatti, a RCS (Rizzoli-Corriere della Sera) è stato concesso il rifinanziamento del proprio debito, per poi andare a fare un accordo con Cairo, di 352 milioni. Non è vero, allora, che le banche non possono concedere credito, ma è vero che banche concedono credito agli amici degli amici e che poi, quando fanno dei danni, come è successo, a pagare è il risparmiatore, perché la truffa delle quattro banche create da voi con la messa in liquidazione è derivata dal concedere concedere finanziamenti che si sapeva benissimo non sarebbero rientrati. Smettetela di raccontare balle al popolo italiano perché veramente i cittadini fuori sono stanchi e chi è stato truffato - ripeto, da voi e della male gestione delle banche italiane - ha perso i risparmi di una vita. È verissimo che un soggetto si è già suicidato e non vorrei accadesse ancora. Analizziamo il testo. Con l'articolo 1 istituite il pegno non possessorio, ossia la possibilità - voi dite per l'impresa, noi diciamo a vantaggio accedere al credito, ponendo a garanzia un bene strumentale dell'azienda, potendo però continuare ad utilizzarlo. in caso di manifestarsi dell'inadempimento, che è comunque stabilito dalla banca stessa, la vendita, l'escussione o l'appropriazione del bene non seguiranno le normali procedure esecutive, pregiudicando quindi la possibilità del debitore di appellarsi e fare opposizione. Quindi questo è un favore bello grosso alle banche, che concederanno credito solo a chi è talmente messo male economicamente che sarà disposto anche a mettere a repentaglio la propria azienda pur di continuare la propria attività: fregato due volte. Che dire poi dell'articolo 2? Introducete nel nostro ordinamento il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di un bene immobile sospensivamente condizionato, ossia il patto marciano, che consente al creditore di soddisfarsi sulla cosa data in garanzia acquisendola o vendendola direttamente al verificarsi dell'inadempimento. Il patto marciano, che si distingue dal patto commissorio, vietato dall'articolo 2744 del codice civile, è per la Cassazione ammissibile solo se non sussiste sproporzione tra l'entità del debito e il valore del bene dato in garanzia, se la vendita o l'acquisizione del bene dato in garanzia avviene sulla base di una perizia di stima, e se prevede l'obbligo per il creditore di restituire al debitore l'importo che eccede l'ammontare del credito. In questo provvedimento, invece, manca la previsione per cui l'erogazione del finanziamento non possa essere condizionata alla presenza di tale clausola, perché non avete voluto inserirla, e considerato il maggior potere contrattuale delle banche, che voi avete fornito e continuate a fornire, questo provvedimento farà sì che gli imprenditori saranno di fatto obbligati ad accettare di fatto il patto marciano, se vorranno continuare la propria attività, e quindi a pagare le tasse. Ve lo ripeterò fino allo sfinimento: di quelle entrate da cui derivano i nostri stipendi, non dimenticavelo mai, perché più voi diminuite le entrate fiscali e meno soldi abbiamo anche per gli stipendi. Manca il Manca il riferimento esplicito al fatto che non debba sussistere una sproporzione tra l'ammontare del finanziamento e il valore del bene immobile dato in garanzia: non l'avete voluto scrivere. Manca il riferimento al fatto che il trasferimento del bene estingue comunque l'obbligazione del debitore, anche se il valore di stima dell'immobile è inferiore all'ammontare del debito residuo. Ora vi chiedo: se l'economia italiana è in crisi, e quindi c'è una svalutazione degli immobili, secondo voi potrà accadere che il bene posto in garanzia sia minore del debito residuo? È possibile, ma voi non avete voluto inserire questa clausola,

Poi, come inadempimento viene definito il mancato pagamento di tre rate non consecutive, se mensili, oppure di una rata se la rateizzazione è superiore al mese. In Commissione il sottosegretario Baretta ha spiegato che se una rata viene comunque pagata, non viene considerato mancato pagamento. Vorrei ricordare che il testo unico bancario definisce come mancato pagamento quella rata che viene pagata oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza, quindi si poteva scrivere benissimo questa spiegazione; invece non avere spiegato che comunque il pagamento della rata va a non costituire inadempimento darà luogo a contestazioni, ma il debitore sì vedrà comunque togliere il bene posto in garanzia. Sempre a favore delle banche. Per non dire di tutte le altre cose che avete fatto con la modifica della normativa sul fallimento. Che dire poi del rimborso ai risparmiatori? Intanto, è un indennizzo, e già utilizzare la parola indennizzo significa che c'è stato un danno. Avete messo dei paletti, che sono i paletti imposti dall'Europa, ma non avete assolutamente spiegato alcune cose e vi sottopongo un dubbio:

sicuramente non avrà la tassazione dell'indennizzo, ma si porrà il problema per l'imprenditore individuale, per l'agricoltore e anche per il coltivatore diretto. auguro che questo dubbio venga risolto in Commissione con la risposta alla nostra interrogazione. Vorrei poi ricordare che tutta la truffa delle quattro banche risulta anche da MiFID sbagliate, che sono compilate a caso. Diverso tempo fa noi abbiamo chiesto le dimissioni di Vegas e ultimamente la trasmissione «Report» ha riportato un documento in cui si dimostra che Vegas ha tolto dalle informazioni il foglio in cui si indica la probabilità di un investimento. Sicuramente noi non daremo la fiducia a questo Governo, che continua a favorire le grandi imprese e i grandi gruppi bancari, e ci auguriamo che i cittadini in tutte le piazze continuino ad urlarvi il loro no, perché è veramente ora che voi andiate a casa.

la prima (articoli da 1 a 3), che prevede l'introduzione di nuovi istituti o la modifica sostanziale di precedenti; la seconda (articoli 4 e 5), modifica, anche in modo sostanziale, le disposizioni previste dal codice di procedura civile in tema di espropriazione forzata allo scopo di rendere le procedure più incisive e soprattutto più rapide; la terza (articolo 6), dove vengono modificate le norme della legge fallimentare, anche in questo caso per accelerarne l'*iter*; la quarta (articoli 8, 9 e 10), forse quella di maggior preminenza e comunque di notevole impatto sociale, che prevede il ricorso al Fondo di solidarietà per l'erogazione di un indennizzo forfettario, nella misura dell'80 per cento di quanto pagato

tenendo conto che l'arbitrato potrà avere anche esito negativo o con risarcimento inferiore al *quantum* forfettario previsto dalla norma. Da ultimo, l'articolo 11 tende a risolvere le problematiche sollevate dalla Commissione europea in ordine alla facoltà, concessa con precedente norma, alle aziende e in primo luogo alle banche, di monetizzare le imposte attive anticipate iscritte in bilancio mediante la loro conversione in credito d'imposta, che, come è noto, sono immediatamente utilizzabili o cedibili. A tale scopo si è stabilito che questo beneficio, per non essere classificato in sede europea quale "aiuto di Stato", sia soggetto al pagamento di un canone annuo sino al 2029. Si tratta di una norma di una complessità - mi sia consentito - astrale che prevede, per la determinazione del canone dovuto una serie infinita di calcoli. La discussione in Commissione finanze è stata ampia e articolata, ma caratterizzata comunque dalla fretta del Governo di definire al più presto il provvedimento. Desidero qui ringraziare tutti i componenti della Commissione e i suoi funzionari per l'impegno profuso. Per quanto concerne gli articoli 1 e 2, viene istituito, all'articolo 2, il cosiddetto patto marciano. Su tale argomento mi sia consentita una breve digressione, perché, al di fuori ovviamente di questa Assemblea, non ci sia chi, novello Don Abbondio, si chieda "Marciano chi era costui?". Elio Marciano era un giurista vissuto ai tempi dell'imperatore Caracalla e, quindi, tra il II e il III secolo dopo Cristo. Secondo gli studiosi di diritto romano, è il primo giurista che abbia posto il fondamentale elemento di diversificazione dal patto commissorio, e cioè quello che preventiva la necessità di una stima del bene pignorato da contrapporre all'ammontare del credito concesso. Le norme di cui all'articolo 1 (pegno mobiliare non possessorio) si applicano unicamente alle imprese, ma perché questa limitazione? Forse i professionisti non necessitano di credito per l'esercizio della loro attività? La possibile apertura in tal senso è stata tuttavia denegata sia dai relatori che dal Governo per motivi che ancora oggi mi sfuggono. Altro appunto è in ordine alle concessioni dell'indennizzo, previsto dagli articoli 8, 9 e 10, ai soli clienti delle quattro banche

da una banca diversa dalle quattro commissariate non deve essere risarcito? Non ha forse subito il medesimo danno? Se la ragione è che nelle quattro banche commissariate vi è stato un input all'acquisto, diciamo non corretto, ci pare che questa ragione non sia sufficiente per escludere dall'indennizzo questa categoria. Inoltre, il risarcimento è limitato - come più volte segnalato in Commissione - ai soli investitori delle quattro banche commissariate e, quindi, non è stato adottato alcun provvedimento a favore dei clienti-sottoscrittori di altre banche - in particolare una di tutta rilevanza situata nel Nord-Est - che hanno acquistato o dovuto acquistare titoli di eguale natura di quelli emessi dalle banche commissariate. Per quanto poi concerne gli istituti di cui agli articoli 1 e 2, essi sono stati strutturati con assoluta posizione di preminenza per il creditore. È pur vero, come sostenuto dai relatori, che sia il pegno non possessorio che il patto marciano si perfezionano con il mutuo consenso, del debitore e del creditore, ma - a mio avviso - ciò non basta. Non può sfuggire che il contraente forte, cioè colui che eroga il credito e quindi le banche, potrebbe "spingere" il debitore a sottoscrivere il patto proponendo interessi e commissioni di basso importo, a fronte della possibilità (reale) di ottenere con pronto effetto la soddisfazione del proprio credito nell'ipotesi di inadempimento. Purtroppo la maggior parte degli emendamenti tendenti alla parificazione delle posizioni è stata respinta. Quali considerazioni finali? Il giudizio sul provvedimento non può essere del tutto negativo, soprattutto per la parte che prevede l'indennizzo dei risparmiatori raggirati, ma - ripeto - solo ad una parte di essi.

fatto ancor più rilevante - a parità di condizione, indennizzi a favore di risparmiatori che hanno sottoscritto i titoli presso altri istituti, con possibile declaratoria in sede di contenzioso di norme in contrasto con i principi costituzionali. a fronte di una pluralità di emendamenti volti a chiarire che l'indennizzo/risarcimento non è soggetto a IRPEF, il Governo si è riservato di decidere su tale argomento, visto l'orientamento negativo del Ministero

Non può sfuggire che sottoporre a IRPEF il risarcimento comporterebbe una non indifferente diminuzione di esso, tale da risultare inferiore all'80 per cento Da ultimo, si ritiene deprecabile il continuo uso della fiducia per l'approvazione di provvedimenti così complessi, in particolare se proposti con decreto-legge e - come detto - di notevole impatto sociale. Una discussione in Assemblea, con tempi non condizionati, avrebbe sicuramente migliorato il provvedimento. Per tutti questi motivi, il Gruppo Forza Italia voterà contro il provvedimento.

del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: